link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

trova origine nel calo di adesioni alle vaccinazioni ed è un atto - lo dico in modo chiaro - di grande responsabilità da parte del Governo e del Parlamento, un atto di responsabilità, di presa in cura e di difesa di di difesa di un diritto costituzionale quale il diritto alla salute. È un provvedimento che nel suo passaggio parlamentare ha impegnato per oltre un mese la Commissione sanità in importanti audizioni e che ha prodotto, proprio a partire dalle audizioni, miglioramenti importanti nel testo approdato in Aula.

contempo accanto all'obbligatorietà dei vaccini, attraverso la modulazione della verifica triennale su un gruppo di vaccini, abbiamo lavorato e lavoreremo ancora per l'adesione consapevole alle vaccinazioni stesse. Abbiamo, altresì,

tenendo insieme il diritto all'istruzione e quindi l'accesso alla scuola. Nel contempo abbiamo rafforzato il percorso di informazione e formazione di tutto il personale sanitario e scolastico sulla vaccinazione. Ciò è importante, perché vuol dire che ci stiamo dotando di una modalità basata sull'informazione e formazione che renda tutti gli operatori capaci di una presa in carico individualizzata e personalizzata

profondamente importante e migliorato, mi colpisce molto che i contenuti del dibattito che lo accompagnano in questo Parlamento siano rivelatori dei limiti e dei pericoli espressi da atteggiamenti di forze politiche

di una stessa medaglia. Lo dico in modo molto chiaro: ho la certezza che gli stessi che oggi usano l'argomento della contrapposizione della libertà individuale sono quelli che, quando parlavamo di unioni civili e del diritto di scegliere in modo libero chi amare,

Viene, per esempio, messo in discussione il valore della scienza, l'autonomia tra scienza e politica. È invece bene ricordare che la scienza e la libertà della ricerca scientifica sono il motore dello sviluppo della società oggi più che mai va detto in modo molto chiaro che la scienza è il primo forte antidoto ai venti della demagogia. Purtroppo siamo in un Paese che sconta la scarsa formazione alla scienza, cioè alle valutazioni comprovate e ripetibili rispetto alle opinioni indimostrate

superiore di sanità e avvalendosi di una commissione tecnico-scientifica integrata in modo specifico da esperti indipendenti e privi di conflitti di interessi, dovrà trasmettere ogni anno al Parlamento una relazione sui risultati della farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali sia stata confermata un'associazione con i vaccini. Vorrei anche dire che da una ricerca del Centro

anche a questo troviamo una risposta importante. Infatti, la consapevolezza dell'importanza dell'informazione e della formazione di tutti coloro che si trovano ad impattare sul tema della vaccinazione,

Siamo infatti convinti che il tema dell'accompagnamento dei genitori per rispondere ai loro dubbi, alle loro domande e al loro diritto di sapere, di essere certi della sicurezza, trovi risposta anche in un altro importante elemento di novità introdotto dal lavoro parlamentare. Mi riferisco all'assegnazione ai consultori della competenza di sostenere la genitorialità, quindi anche del tema della prevenzione e della cultura della vaccinazione fin

che anche l'Italia ha sottoscritto ma non sempre praticato, sono soggetti di diritto autonomi e in questo caso sono titolari del diritto alla salute, che viene esercitato tramite i genitori che ne sono i legali rappresentanti. Sia chiaro però che i genitori non sono liberi di decidere della salute di un bambino come cosa loro, ma devono rispettare il principio del superiore interesse del bambino stesso, senza che su di esso prevalgano scelte od opinioni personali. Ricordo che nel 2014 la patria potestà è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale. Questa responsabilità genitoriale va aiutata e accompagnata esattamente attraverso questo passaggio di formazione e informazione e questa presa in carico individualizzata, a partire da un percorso che rassicuri i genitori sulla certezza delle cure, ricordando che i vaccini sono ad oggi il farmaco più sicuro. Quindi il tema è esattamente questo: sostenere il diritto alla salute e avere un dibattito, anche all'interno di questo di questo Parlamento, basato sulle evidenze scientifiche e non sulle credenze popolari. E la politica è esattamente questo: riconoscere, valutare e sostenere il diritto alla salute, che è un diritto individuale e un diritto collettivo, soprattutto in un momento nel quale viviamo Grazie a una responsabilità collettiva, perché solo se c'è coesione sociale, solo se questi due aspetti convivono, potremo essere capaci di rispondere ai mille problemi di questo nostro Paese.

il dibattito sul decreto-legge in conversione sulle vaccinazioni risente di una inopinabile, stucchevole e preconcetta manipolazione

Le vaccinazioni non hanno, né devono, né possono avere il colore di un partito o di un movimento, di una parte o dell'altra. Non appartengono all'uno, né appartengono all'altro. Sono una grande conquista scientifica per il bene salute di ogni singola persona e della comunità. Ricorrono in questo tempo, permeato di *fake news*, definite anche le "camere dell'eco" o le "bolle informative", dove a qualcuno che grida tanti ingenuamente seguono e fanno eco, interrogativi sorprendenti, direi anche fortemente preoccupanti, fino a un'affermazione di tale fatta: è meglio evitare le vaccinazioni. Risulta evidente che il contrapporsi alle vaccinazioni è diventata per alcuni, e temo negli ultimi tempi ingenuamente per tanti, una bandiera dalle tinte fosche e con idee poche e confuse, nonché del tutto fuorvianti. Rilevo che bene si è fatto, nel corso della discussione che ha caratterizzato i lavori della 12ª Commissione, a sottolineare ripetutamente che il decreto-legge ha un suo fondamento scientifico e che, tramite la responsabilità politica del Senato ora e della Camera successivamente, necessita di una rapida conversione in legge. Il tema vaccinazioni è scientifico, ancor prima di tutto. L'alto livello di copertura vaccinale osservato in Italia fino al 2012 per le vaccinazioni oggetto di programmi nazionali o di diffusi programmi regionali e in maniera più evidente per le vaccinazioni obbligatorie ha determinato un significativo decremento dell'incidenza delle malattie prevenibili da vaccinazione. E sottolineo "significativo decremento", che ha un peso di argomentazione scientifica. Pertanto richiede indispensabili competenze e rigorose argomentazioni, per il vero caratteristiche queste che dovrebbero comunque sempre essere la guida in un dibattito politico. Una politica senza una cultura specifica di base, senza consapevolezza e rigore dei fondamenti si trasforma in vuota e pericolosa propaganda; pericolosa sia perché inquina il dibattito, sia perché finisce con il vanificare il riconoscimento di un diritto fondamentale. E la salute è un diritto fondamentale. Nel dibattito sull'obbligatorietà delle vaccinazioni vengono richiamati due diritti, quello alla salute e quello all'istruzione, entrambi garantiti dalla Costituzione; pur tuttavia, questi due diritti hanno una diversa portata. All'articolo 34 della Costituzione viene sancito

per il lavoro svolto, in sintonia, in collaborazione, con pacatezza di obiettivi e con rigore argomentativo, dalla Commissione igiene e sanità e con il Governo, rappresentato dalla ministra Lorenzin, finalizzato alla mitigazione delle sanzioni, anche con l'approvazione di un emendamento di cui sono firmatario. Altro, forse ancor meglio definirlo previo e preliminare, è il diritto alla salute. Nell'ordinamento italiano esso è riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Il diritto alla salute è riconducibile, in ambito quindi squisitamente giuridico, alla categoria dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della Costituzione,

poiché rende possibile il godimento dei diritti di libertà. Detto in una maniera più mediaticamente percepibile, non c'è libertà se non c'è riconoscimento della vita; è il valore previo, quello della vita, che ci dà la possibilità di poter realizzare qualsiasi altro diritto. La salute, quindi, rappresenta non solo un diritto primario dell'individuo, ma è anche interesse preminente della collettività. Infatti, a tal fine sono previsti sia interventi diretti alla cura sia alla prevenzione delle malattie. È in questa cornice costituzionale che si inscrivono le vaccinazioni, appunto come diritto nonché dovere nell'interesse dell'individuo e della collettività nella prevenzione primaria delle malattie. prevenzione primaria delle malattie. Tale prevenzione, a cui ci si richiama attraverso le vaccinazioni, consiste in un insieme di interventi volti a favorire e mantenere lo stato di benessere ed evitare l'insorgere di malattie, a livello di singolo individuo, di collettività e di ambiente. gli obiettivi del decreto-legge sono specificamente orientati a dare una risposta a quattro di questi punti: proteggere il singolo; controllare le malattie nella popolazione; circoscrivere le malattie; e, possibilmente, eradicarle. Le vaccinazioni proteggono da malattie gravi e rappresentano uno degli interventi più efficaci e sicuri in sanità pubblica.

che, per eminenti ricercatori, scienziati, storici della medicina e per tutti, rappresentano uno dei segni più tangibili del progresso della medicina insieme agli antibiotici. Grazie alle vaccinazioni, l'incidenza di molte gravi malattie è drasticamente diminuita. Ma se non vengono mantenute coperture vaccinali ottimali, alcune malattie eliminate o diventate rare possono rapidamente riapparire, perché gli agenti infettivi che le causano continuano a circolare in tutto il mondo. Oltre alla riduzione della mortalità e della morbilità correlate alle malattie infettive evitate, l'efficacia delle vaccinazioni è evidente anche in termini di riduzione della spesa sanitaria. Se una vaccinazione, così contemplata, richiede circa 15 euro a persona, la somma che dovrebbe essere messa a disposizione per insorgenza della malattia è di gran lunga superiore ai 15 euro a persona. persona. In Italia tutti i livelli di copertura vaccinale per malattie ad alta contagiosità sono attualmente al di sotto dello *standard* accettabile del 95 Basti richiamare la copertura vaccinale più bassa, che si riferisce alla vaccinazione contro la varicella, pari ad appena il 46,1 per cento, mentre la maggioranza di tutte non raggiunge nemmeno il 95 Dire che bisogna ricorrere all'obbligatorietà vaccinale solo in caso di epidemia non solo è molto grave, ma - lasciatemi usare un'espressione che può sembrare forte in quest'Assemblea - significa ignorare del tutto i fondamenti del significato della vaccinazione.

che hanno alzato la bandiera del no vax. Queste persone devono sapere in maniera molto, ma molto seria che sulla loro pelle e sul loro non sapere si sta giocando una partita politica che a me e tanti di noi non appartiene assolutamente.

che la migliore immunizzazione sarebbe quella secondaria alla "fisiologica" trasmissione della malattia, senza ricorrere alle vaccinazioni, che risulterebbero pericolose.

il morbillo, nei bambini che contraggono il morbillo vi è una complicanza che si chiama encefalite, che si presenta in un caso ogni mille.

un caso ogni 1.300-2.000 porterà alla cosiddetta panencefalite sclerosante subacuta; per chi non ha conoscenze in merito, credo sia opportuno, prima di fare affermazioni avventate, almeno valutare la letteratura in proposito. mossa un'altra osservazione, che mi ha incuriosito notevolmente e che si riferisce a una Regione d'Italia dove si ritiene che sia anticostituzionale il ricorso all'obbligo di vaccinazione, e che si sia raggiunta già una copertura vaccinale tale e idonea da impedire che si ricorra all'obbligatorietà. Ebbene, la curiosità di chi per tanti anni ha fatto attività di ricerca e di didattica scientifica l'ha indotto a fare una riflessione e ha visto che in quella Regione - avete capito perfettamente che mi riferisco al Veneto ci sono stati, da gennaio a tutt'oggi, 200 casi di morbillo, su una popolazione *in toto* di 5 milioni di abitanti.

il 97 per cento di copertura vaccinale, non obbligatoria (perché hanno una maturità tale da non aver bisogno della obbligatorietà per vaccinarsi); indovinate e date un numero a caso di quanti casi di morbillo ci sono stati: con il doppio della popolazione, da gennaio 2017 a fine giugno 2017 vi Che cosa può significare tutto questo? Significa che la dimensione della obbligatorietà evidentemente va a supplire una carenza riconducibile a una mancata copertura vaccinale, laddove non c'era la obbligatorietà, ma solo la consigliabilità della vaccinazione. Questo provvedimento, quindi, ha una sua eticità di ordine sociale e un suo fondamento di ordine scientifico. Ho sentito anche qualche dato nella discussione di ieri di ieri sui casi di morbillo risalenti al 27 maggio 2017; forse è meglio aggiornarsi quando si interviene in Aula su determinati argomenti.

chi dice che l'obbligatorietà non risponde a criteri di eticità si deve assumere la responsabilità di questi decessi. Ma poi ci sono anche, come dicevo prima, le cosiddette bolle informative, una sorta di *fake* *news*, che

Si dice che un miglioramento delle misure igieniche e sanitarie eradicherà le malattie e quindi che i vaccini non sono necessari. Assolutamente falso; se fosse così semplice basterebbe ricorrere alle più elementari norme igieniche e non ci sarebbe più la trasmissione di virus e di batteri. Forse qualche piccolo studio nell'ambito dell'infettivologia e della microbiologia credo sia opportuno farlo. Se così avessimo risolto tutti i problemi avremmo trovato la panacea di tantissime patologie. Altra falsa notizia: i vaccini si associano a parecchi effetti dannosi a lungo termine, ancora sconosciuti, le vaccinazioni possono essere anche fatali. C'è una contraddizione in termini: si dice che possono essere legati a eventuali effetti negativi, che non sono conosciuti, ma, in quanto inconoscibili e non prevedibili, perdono di per sé la loro sostanza di ordine argomentativo. Se non sono conoscibili, fatemi capire quali possono essere gli effetti che si possono determinare. Non entro nel particolare perché evidentemente il tempo a disposizione non mi consente di affrontare nello specifico le singole tematiche. Vado rapidamente a citare altre false notizie. Si dice che il vaccino combinato contro difterite, tetano e pertosse e quello contro l'epatite sarebbero responsabili della sindrome della morte in culla, ma non è assolutamente vero: non c'è una ricerca scientifica che li ponga in

senza specificare che all'interno di qualsiasi composizione farmaceutica ci sono eccipienti, additivi e altre sostanze, che non starei qui ad indicare e che sono necessari per la loro produzione.

contestare che non è sufficiente quello che sto dicendo. Ebbene, gli studi condotti non hanno mai dimostrato l'esistenza di una correlazione causale tra vaccini contenenti mercurio e autismo

Potrei continuare ancora, perché in questi giorni, purtroppo, drammaticamente, tante *fake news* vengono lanciate, supportate da pseudo-pubblicazioni scientifiche

Signor Ministro, signori senatori, voglio ringraziare ancora, per il lavoro svolto nell'ambito della Commissione Igiene e sanità, la presidente De Biasi, la relatrice senatrice Manassero, lei, signor Ministro, e tutti coloro che hanno collaborato con grande sobrietà,

credo che l'aspetto più significativo, che nessuno può negare, è che un genitore per il proprio figlio vuole il meglio. Avete trasformato il buonsenso,

Credo ci siano due principi nella ricerca e nella medicina. Il primo principio è quello socratico, per cui io so di non sapere; la ricerca parte sempre da questo presupposto e qualunque posizione autoreferenziale porta al fallimento della ricerca. L'altro principio della medicina è che ogni individuo ha una specificità. Ogni individuo, soprattutto ogni bambino, ha diritto a un'attenzione specifica e individuale.

alla specificità della salute di ogni bambino e, quindi, al rispetto di chi se ne prende cura. È un modo brutale di sostituirsi ai genitori, degno di un qualche passato ventennio, ed è da rigettare. Quello che ho sentito in quest'Aula, l'alleanza medico-paziente che è stata invocata (e che casualmente viene sempre invocata quando si vuole rigettare sul paziente la responsabilità della sua cura in termini di spesa), qui viene qui viene negata. È un'impostazione arrogante quella che viene stabilita da un Governo che pretenderebbe di avere l'autorevolezza e la credibilità per farlo, ma evidentemente non le ha

tutto il danno che deriva dall'aumento del contenzioso e vorrei che ci si ricordasse poi da dove ha avuto origine il contenzioso. Ha avuto origine anche da questo.

abbiamo assistito al potere di veto che viene consentito alla Commissione bilancio. La Commissione bilancio ha mostrato un atteggiamento molto particolare rispetto al provvedimento al nostro

senza alcun trasparenza. Quando si pone il veto per eccesso di spesa su una proposta di riduzione del numero di vaccinazioni obbligatorie si perde, infatti, ogni credibilità.

la relatrice a chiedere la modifica del titolo. Spero che avremo la possibilità, in sede di esame degli emendamenti, di entrare anche nel merito di queste particolarità che sono state previste nel provvedimento.

un anno di reddito di cittadinanza per risanare due delle numerose banche che voi avete spolpato. Detto questo, entriamo nel merito, per dire che ci sono voluti diciassette giorni tra l'annuncio del decreto-legge e la sua giorni durante i quali ci si immagina che il decreto sia stato valutato, soppesato, perfezionato, reso impeccabile. Invece, nulla di tutto ciò. In Commissione arriva un testo, del quale si discute, si approfondiscono temi si approvano emendamenti. Intanto, arriva un emendamento del relatore che riscrive l'articolo 1, che è il cuore del provvedimento; ma non è ancora a punto, e lo si subemenda. Poi ne arrivano altri e la storia si ripete più volte. L'ultimo emendamento del relatore è datato lunedì sera, ultima seduta della Commissione, e di questo noi stiamo discutendo. Dopodiché, apprendiamo che la Commissione bilancio non ha approvato alcuni emendamenti inseriti in quel testo. Quindi, tutti noi stiamo discutendo di un testo che non è quello su cui poi dovremo ragionare relativamente agli emendamenti che poi presenteremo in Aula. Durante questo periodo, però, gli scienziati che consigliano il Ministro si convincono che dodici vaccini obbligatori sono troppi. Si passa a dieci. Forse perché, nottetempo, la scienza è cambiata? Caspita, che scoperte repentine! Contemporaneamente, si aggiungono quattro vaccinazioni raccomandate, di cui due sono quelle che prima erano obbligatorie. Cosa mai avranno scoperto questi scienziati per declassarli da obbligatori a raccomandati? La riduzione da dodici a dieci vaccini obbligatori dimostra che ciò che era stato propagandato come assoluto, come scienza, per il bene dei bambini diventa relativo; allora perché non nove, otto o sette vaccini? Signor Sottosegretario, io sono curioso. Ho provato a cercare questa risposta, ma non l'ho trovata. Sottosegretario, io sono un medico ed il medico è il primo che deve dare risposte ai cittadini che consiglia di vaccinare. Io ci metto la faccia, ma lei mi deve dare risposte convincenti; altrimenti, la faccia con quei genitori ce la metta lei! Ritengo che il provvedimento uscito dalla Commissione sia profondamente sbagliato nella sua impostazione generale, in quanto in ambito sanitario è indispensabile che i due elementi (individuo, da un lato, e salute pubblica, dall'altro) si incontrino sullo stesso piano senza che uno prevarichi sull'altro. Il diritto della persona e l'interesse generale sono compatibili e sta al Governo trovare un giusto equilibrio. In questo caso, la scelta del Governo è di imporre le vaccinazioni, visto che non è in grado di muoversi per trovare il giusto equilibrio di questa società complessa. Cerca la via breve, mettendosi contro la società stessa con la scusa di proteggere il singolo. Questo metodo è completamente sbagliato, come evidenziato dalla più recente letteratura, la famosa medicina basata sull'evidenza. La meta-analisi Cochrane del 2017 del 2017 analizza trentotto pubblicazioni internazionali e raccoglie le opinioni e le esperienze dei genitori a proposito delle informazioni fornite al momento della vaccinazione infantile routinaria: sono il modo e le parole con cui vengono comunicate le informazioni a influenzare le decisioni dei genitori in materia di vaccinazione infantile. I genitori vogliono essere informati per tempo. Vogliono trovare personale sanitario disponibile e preparato in grado di rispondere ai loro dubbi e alle loro paure. Un personale sanitario disponibile a discussioni aperte e rispettose con loro, in modo attento, sensibile, non giudicante, creando un ambiente favorevole al processo decisionale. Si aspettano che il personale sanitario abbia a cuore l'interesse del bambino e che non sia guidato da incentivi finanziari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In sostanza, il genitore bene informato da un professionista credibile accetta il consiglio o, meglio, la raccomandazione alla vaccinazione. L'obbligo allontana la vaccinazione e questa è medicina basata sull'evidenza. Pertanto, bisogna lavorare molto sulla credibilità e sull'autorevolezza, sia dei professionisti sanitari sia delle istituzioni, cosa che questo decreto non fa. Questo decreto non mette risorse nel mondo sanitario. Avete demolito i distretti e in certi ambiti le vaccinazioni si concentrano in poche ore, con cadenza mensile o bimestrale, spesso in luoghi fatiscenti, con carichi di lavoro che non consentono quel dialogo. Di fronte a un genitore preoccupato, anziché prenderlo per mano e accompagnarlo in un percorso difficile ma rassicurante, perché si attui quell'alleanza terapeutica tra il cittadino e le istituzioni, voi che fate? Obbligate all'assunzione di una procedura, pena la non iscrizione alla scuola dell'infanzia e sanzionate amministrativamente con 3.500 euro di multa, la qualcosa creerà decine di ricorsi ai tribunali, intasandoli. Questo decreto-legge lascia aperti molti spazi nei quali gli avvocati possono inserirsi, dilatando i tempi e consentendo, tra l'altro, ai genitori di spendere meno delle multe che voi sanzionate. Quindi, oltre al danno la beffa: non avremo copertura vaccinale e avremo i tribunali intasati. Veramente geniale! Questa ottusità di comportamento ha indotto a negare ai cittadini legittime richieste, come la rimodulazione dello schema esecutivo delle vaccinazioni. Perché non spostare la vaccinazione della rosolia alle sole ragazze in età adolescenziale? Questa domanda l'ho rivolta a diversi esperti in Commissione durante le audizioni ma nessuno mi ha risposto. Si parla di medicina personalizzata, ma non per la somministrazione dei vaccini. interessante notare come entro il 10 settembre di quest'anno i genitori dovranno presentare a scuola la documentazione delle avvenute vaccinazioni, mentre dall'anno 2019-2020 il sistema sarà semplificato (parola di grande effetto, ma dal significato opposto quando scritta in una norma). Perché non graduare nel tempo l'applicazione? Mi riferisco a un emendamento che è stato bocciato dalla Commissione bilancio. Vorrei sottolineare quale sia l'attenzione che questo Governo ha nei confronti dei bimbi non vaccinati: chiede a tutto il personale sanitario e scolastico di presentare idonea certificazione circa lo stato vaccinale al medico competente della struttura, che valuterà come e se immunizzare in base alla legge n. 81 del 2008 a tutela del lavoratore e conseguentemente e indirettamente dei bimbi.

avete dovuto escogitare il blocco scolastico. Ed ecco, quindi, che, a fronte di un maggior lavoro degli operatori, si sono trovati un po' di fondi, spostandoli però dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Mi verrebbe da dire: così avremo figli un po' meno istruiti, ma vaccinati. Comunque, tranquilli, perché il Governo ha pensato alle iniziative per informare sia il personale della scuola sia gli alunni, stanziando l'incredibile cifra di 200.000 euro. Concludo dicendo che è il momento che il cittadino sia rimesso al centro. L'ho già scritto nella mozione sugli *screening*: bisogna incentivare il cittadino disciplinato, quello che rispetta le regole, che crede nel sociale e accetta un rischio, seppur piccolo, per una visione sociale;

i colleghi della Commissione sanità, la relatrice Manassero, la Presidente della Commissione e ovviamente il Governo per il lavoro davvero approfondito che è stato fatto in queste ultime settimane in Commissione sanità nella nell'approfondimento, nello sviscerare davvero in maniera incredibile il provvedimento che oggi stiamo esaminando.

a numerosissime audizioni che hanno visto la presenza di rappresentanti della scienza, delle istituzioni, delle associazioni dei cittadini e dei genitori (quelli favorevoli ai vaccini e quelli

del provvedimento che il Governo ha adottato in un momento difficile, di urgenza, che non è stata dichiarata da una improvvisa valutazione di qualcuno, ma che è stata e viene sollecitata ormai da più di tre anni dall'Organizzazione mondiale della sanità, perché lo stato lo stato delle vaccinazioni in Italia è estremamente preoccupante. Non voglio ripetere l'elenco delle questioni, i dati statistici e i numeri, che sono stati

che, in realtà, da parte di qualcuno, si sia trasformata in guerra la necessità di rivedere e aggiornare la profilassi, che è un'altra cosa.

infatti permetterci di avere opinioni, di chiedere cambiamenti, di condurre battaglie per le nostre opinioni,

hanno la responsabilità di offrire ai cittadini italiani delle verità scientifiche. Noi non abbiamo questa responsabilità e questa capacità e non possiamo e non possiamo avere l'arroganza di assumercele. Dopodiché, nella discussione che abbiamo aperto non solo nei luoghi istituzionali, ma anche nei luoghi che ci hanno visto partecipare a confronti con i cittadini, abbiamo condiviso la giustezza di alcune modificazioni, migliorando il decreto-legge, che è intervenuto su questioni cui la politica è chiamata a dare una risposta e e non sull'interpretazione scientifica. Vorrei ricordare a tutti che sull'urgenza e sulla necessità c'è

l'indicazione che viene data da autorevoli istituzioni di Paesi stranieri sia quella di non venire in Italia perché c'è il pericolo di epidemie di morbillo, e non solo.

degli eventi avversi che possono accadere quando ci si vaccina, ma che possono accadere anche se prendiamo un antidolorifico o se facciamo una puntura perché abbiamo un dolore alla schiena. Purtroppo ciò può accadere. In questo provvedimento abbiamo chiesto però che ci sia una maggiore trasparenza anche rispetto al tema degli eventi avversi, ma questo non può essere, esattamente come dicevo prima, l'elemento che ci può portare a ignorare l'importanza e la necessità della cosiddetta copertura di gregge, di cui il nostro Paese in questo momento ha necessità e urgenza.

un elemento di negatività e rappresenta il dissenso di una parte dei cittadini italiani (che è una minoranza per la quale sono preoccupata)

ho sentito parlare poco del numero enorme di famiglie e genitori che ci chiedono di approvare presto il provvedimento perché i loro figli, che hanno patologie molto serie e non possono essere sottoposti a vaccinazioni, vivono una condizione di vita di isolamento. Non possono andare a scuola, non possono avere possibilità di relazioni sociali e crescono in un isolamento relazionale che certamente non fa bene a quei bambini e alla nostra società. Di queste famiglie e di questi bambini abbiamo parlato pochissimo. Credo che di loro dovremmo invece parlare e che nei loro confronti dovremmo assumerci una delle

ha avuto l'opportunità, per la prima volta, di potersi vaccinare contro la poliomielite. Anche io era una bimbetta in quegli anni e, purtroppo,

alla malattia che colpì una mia amichetta di giochi. Venti giorni dopo questo evento doloroso che aveva portato quella famiglia nel dramma, nel paesello dove vivevo e crescevo arrivò l'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione antipoliomielitica, che allora era - se non erro - il vaccino Salk ed era a pagamento, cosa che quindi non consentiva a

la reazione della mia mamma che, di fronte all'opportunità di potersi permettere la vaccinazione per la propria figlia, sembrava aver conquistato davvero il mondo.

di non attribuire al provvedimento responsabilità che non ha e, cioè, quella di voler allontanare con l'obbligo vaccinale dalle vaccinazioni. È il contrario. È vero che ognuno di noi avrebbe preferito che in Italia non si arrivasse ad un livello

voluto che la copertura vaccinale fosse la risposta spontanea di adesione dei cittadini. Non è stato

un'informazione puntuale e una verifica costante dei dati vaccinali nel corso dell'anno e che il Parlamento venga informato in questo senso. Abbiamo responsabilmente migliorato questo provvedimento per tutta la parte riguardante

al ragionamento che si sta facendo sul dramma del grande sovraffaticamento di pratiche e di percorsi burocratici cui i cittadini verrebbero sottoposti per corrispondere a questo obbligo,

per rendere assolutamente trasmissibile per via telematica tra i due soggetti istituzionali tutto quanto riguarda l'adesione e lo stato vaccinale dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno la scuola. quindi che questo serva anche a richiamare a una maggior responsabilità organizzativa le nostre istituzioni che, quando vogliono,

a quello che viene definito da parte di tutti uno dei fattori più importanti in medicina, e cioè la prevenzione. Ricordo che lo stesso Ministro, parlando di prevenzione durante la trattazione

la necessità di rinnovare le attrezzature all'interno degli ospedali e di rivedere il loro apparato edilizio. La prevenzione, a detta del Ministro, riguardava

seguente:« La promozione della salute e la tutela del benessere psicofisico della persona richiedono strategie intersettoriali e trasversali nelle quali siano coinvolte le istituzioni centrali e locali e la società civile.

indovinato - movimenti migratori che stanno interessando il Paese e che richiedono specifiche azioni per la tutela della salute individuale e collettiva. D'altro canto, si potrebbero ulteriormente accentuare si potrebbero ulteriormente accentuare le azioni di disturbo dei gruppi anti-vaccinisti nei confronti dell'azione di governo che mira al consolidamento delle coperture vaccinali, anche in considerazione dell'afflusso migratorio citato, spesso da zone dove il sistema sanitario non è riuscito a garantire tassi vaccinali adeguati». detto il Ministero della salute nella direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione nel 2016. Il Ministero, pertanto, aveva piena consapevolezza di quello che sarebbe successo non solo

lo stesso Ministero rendeva necessaria l'attività di comunicazione e informazione istituzionale, avendo questa un ruolo strategico in tema di salute, in quanto finalizzata a rafforzare una migliore conoscenza, una maggiore consapevolezza della popolazione, in generale, e a favorire, più in particolare, l'adozione di stili di vita e di comportamenti salutari. Ora, questo è ciò che è mancato in assoluto da parte del Ministero, da parte della signora Ministro, da parte del Governo. Si propongono delle innovazioni piuttosto onerose

il Ministero ravvedeva all'interno della propria organizzazione la necessità di fare una campagna di promozione anche sui *social* *forum* oltre che sulla stampa, e la dava come spunto nel 2016, mi chiedo perché

rischi per la popolazione con le nuove vaccinazioni, ma sono altresì certo che basti avere una condivisione circa l'azione di Governo da parte della popolazione, che ha il diritto di essere informata e il Governo ha il dovere di dare le informazioni.

la discussione pubblica che si è prodotta sui vaccini esprime una polarizzazione che sempre più ha trasformato il discorso scientifico in un patteggiamento ideologico, e cioè in una falsa rappresentazione della realtà, un problema - potremmo dire - quasi epistemologico. Da una parte il vaccino è visto dagli antivaccinisti come il risultato di un complotto delle case farmaceutiche e dei poteri forti contro la salute pubblica; dall'altra vi è una campagna mediatica che annuncia il ritorno della peste nera bubbonica per significare e poi giustificare la decretazione d'urgenza e il trattamento sanitario obbligatorio di massa; posizione che però, declinata male e strutturata peggio, ha posto i giusti dalla parte del torto. Il risultato di questo scontro è un grande disorientamento, una grande paura nel corpo sociale, che mina l'informazione consapevole e il diritto alla salute. Che la credibilità della classe politica sia ai minimi storici è noto a tutti. Questa sfiducia, però, colpisce non solo i rappresentanti politici, ma ogni istituzione che sia a essi direttamente o indirettamente collegata. Le istituzioni medico‑sanitarie non fanno eccezione. Se non si crede più al medico, allora, semplificando, si cercano risposte nella Rete con l'illusione di sentire tutte le campane e farsi un facile pensiero proprio. Ma non è così. La Rete è uno strumento universale di facile ed economica accessibilità, ma non è uno strumento democratico e attendibile di informazione, bensì l'esatto contrario, perché settorializza, specializza, indicizza e ripropone esattamente ciò che ognuno di noi vuol farsi sentir dire; praticamente si è portati cognitivamente a dar peso alle notizie che confermano le proprie tesi e i propri pregiudizi. La Rete è piena di *fake news*, spesso profumatamente pagate. Il dibattito in Rete è il campo da gioco di *trolls* e *haters*, dove l'opinione di un *blogger* ha lo stesso peso, spesso maggiore, di chi pubblica su riviste scientifiche. Antivax, freevax, provax, curiosi, convinti, scettici o dubbiosi nel mondo virtuale procedono senza controllo rinforzando le proprie opinioni. Per affrontare la questione vaccini, invece (come quella dell'immigrazione o della sicurezza), bisogna iniziare a dotarsi di strumenti e metodi, che sappiano iniziare a distinguere la percezione della realtà dalla realtà stessa; una questione - come dicevo - epistemologica, perché si tratta di confrontarsi con le basi del sapere. La medicina non è una scienza esatta e, nell'incessante attività di ricerca che la riguarda, non è raro che un nuovo studio smentisca una tesi precedentemente data per certa. Quest'attività viene definita progresso scientifico, ma deve avvenire all'interno della comunità scientifica, cioè deve essere fatta da scienziati, utilizzando i metodi propri della scienza, e i risultati devono essere accreditati da organi ufficiali, quali riviste scientifiche, università e altre istituzioni che ne garantiscano la correttezza. La correttezza non deve essere confusa con l'infallibilità, in quanto è semplicemente l'ammissione che, in un dato momento storico, questa è la frontiera raggiunta dalla scienza. Quando si discute di politiche sanitarie, infatti, non è possibile prescindere da ciò che la scienza è giunta a definire come certo, anche se un giorno verrà smentito o integrato da altre scoperte. È da qui che bisogna partire per qualsiasi confronto; altrimenti il risultato della discussione sarebbe uno scontro tra opinioni che resterebbero irriducibili, insolvibili e inverificabili. E a questo risultato stiamo quasi arrivando.

Nel momento in cui cala l'immunità, io posso ipotizzare che siano facili dei focali epidemici e, quindi, una diffusione dei casi con annesse le complicanze, i costi e la mortalità. un obbligo impostato in modo non corretto, senza un consenso consapevole, non va molto lontano.

Riconosco che tra i casi di morbillo richiamati dall'autorità, con l'obiettivo di sradicarlo - secondo l'Organizzazione mondiale della sanità doveva essere sradicato nel 2015 in Italia nel solo 2014 vi sono stati 1.674 casi, con un'incidenza maggiore registrata proprio nei bambini sotto i cinque anni di età. Per un paziente su tre è stato inoltre necessario il ricovero ospedaliero.

L'Organizzazione mondiale della sanità individua la causa delle ricorrenti epidemie di morbillo proprio nell'aumento del numero dei genitori che non vaccinano i propri figli. L'Istituto superiore di sanità

Sebbene questa possa sembrare una percentuale ancora elevata, in realtà è ancora lontana da quel 95 per cento fissato dal Piano nazionale prevenzione vaccinale. Sotto il 95 per cento, il numero di persone esposte al contagio diventa abbastanza elevato da permettere agli agenti patogeni di diffondersi all'interno della popolazione durante un'epidemia. Scompare, cioè, la famosa immunità di gregge, ossia la protezione di cui godono indirettamente anche i soggetti non immuni, come i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età di vaccinazione, o gli adulti che non hanno mai sviluppato l'immunità. Poiché contro il morbillo viene somministrato il vaccino MPR, che immunizza anche contro la parotite e la rosolia, la copertura nella popolazione risulta inadeguata anche per queste due malattie. I dati più aggiornati mostrano che la copertura vaccinale inizia a restringersi anche per altre malattie infettive. I numeri variano da Regione a Regione, ma nel 2014 le coperture medie nazionali per poliomelite, difterite, tosse ed epatite b sono tutte scese, anche se di poco, al di sotto del 95 L'analisi dell'Istituto superiore di sanità divide la storia recente in due fasi: una prima, dal 2000 al 2012, in cui le coperture si sono mantenute sostanzialmente stabili e, nel caso del vaccino MPR, sono cresciute; una seconda, dal 2012 al 2014, in cui le coperture hanno iniziato a restringersi, soprattutto contro morbillo, parotite e rosolia. Come evidenzia l'Istituto superiore di sanità, i dati del 2014 2014 confermano che il calo registrato a partire dal 2012 non è una flessione temporanea, ma una tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno. Negli ultimi mesi il problema del calo delle coperture vaccinali ha attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, soprattutto in seguito ad alcune notizie: ricordiamo il primo caso nel Paese da trent'anni; la morte per pertosse a Bologna di una neonata non ancora in età di vaccinazione e sette casi di meningite in Toscana.

per la sottocultura delle teorie del complotto. Non è difficile imbattersi in materiale antivaccinista, in siti e in *blog* che trattano di argomenti del genere, dalle verità nascoste, al nuovo ordine mondiale, alla fanta archeologia, alle scie chimiche, alle più diverse tesi alternative alla scienza ufficiale. Tuttavia, le motivazioni alla base della decisione di non ricorrere ai vaccini sono le più diverse e solo una minoranza abbraccia un antivaccinismo militante. I più nutrono timori e dubbi che non riescono ad essere dissipati, perché sono disorientati da informazioni carenti e contraddittorie, anche da parte di alcuni medici. La sensazione di mancata trasparenza provoca sfiducia e sospetto verso le istituzioni sanitarie e genera il bisogno di cercare risposte altrove. C'è poi una difficoltà di cui tener conto, che va al di là della problematica della disinformazione. Come molte altre discussioni su temi scientifici o medici oggetto di controversie sociali, anche quella dei vaccini non è solo una discussione sui vaccini. Fatti ed evidenze possono non riuscire a scalfire le posizioni contrarie, perché queste sono il frutto di esperienze personali, valori morali, convinzioni politiche e pregiudizi. In altri termini, ai fatti si oppongono i *frames*, immagini, schemi interpretativi, cornici di senso, entro cui la realtà viene sistemata e adattata. Ad esempio, se per qualcuno i vaccini rimandano alla medicina ufficiale, o Big Pharma, e se questi elementi sono già inquadrati in un *frame* negativo, allora lo saranno anche i vaccini. Infine, come è stato affermato e ripetuto più volte durante la discussione, i vaccini sono vittime del loro stesso successo. I risultati ottenuti in seguito alle campagne di vaccinazione, dalla scomparsa della poliomelite in Occidente all'eradicazione globale del vaiolo, hanno fatto perdere in poco tempo la memoria delle epidemie del passato, anche quello più recente. Questo induce oggi molti a sottostimare i rischi delle malattie infettive e a sovrastimare quelli dei vaccini. Coinvolgere i cittadini nell'attività di divulgazione potrebbe aiutare a rompere i *frames* negativi e ad allontanare le paure. Nel frattempo, anche dalle Regioni è arrivato l'invito a considerare l'introduzione dell'obbligo di vaccinazione per l'accesso alle scuole e si discute anche del ruolo e della responsabilità degli operatori sanitari e dell'ipotesi di sanzionare i medici che sconsigliano i vaccini; tutte ipotesi che hanno portato, poi, a una sintesi nel decreto-legge in esame. I fatti, però, possono non bastare a modificare i *frames* negativi ma, visti i numerosi luoghi comuni ed errori che circondano l'argomento,

se noi per sicurezza al cento per cento intendiamo la certezza assoluta che la somministrazione di un vaccino comporti un rischio pari a zero, allora questa certezza non esiste, come non esiste per alcun farmaco, terapia, intervento chirurgico e, in generale, direi per qualsiasi attività umana. Del resto, è proprio per questa ragione che si prendono tutte le precauzioni per cercare di abbattere il più possibile i rischi, come avviene - ad esempio - con le procedure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Come per i farmaci, anche per i vaccini la valutazione della sicurezza avviene quando se ne studia l'efficacia, durante le diverse fasi di sperimentazione, e l'intero processo è sottoposto alle leggi e al controllo degli enti regolatori, dell'AIFA e dell'EMA, che solo dopo la fine degli studi autorizzano l'uso e l'immissione in commercio del nuovo vaccino. Ma i controlli proseguono anche dopo l'autorizzazione, attraverso il sistema della sorveglianza, che raccoglie tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse inviate agli operatori sanitari. addietro - ad esempio - l'AIFA ha bloccato in via precauzionale alcuni lotti di vaccino antinfluenzale (il Fluad) dopo la segnalazione di alcune morti sospette. Il divieto è stato poi rimosso, dopo che le analisi hanno escluso qualsiasi legame con i decessi, come confermato anche dall'Agenzia Oltre alla sorveglianza ci sono anche i dati provenienti dagli studi pubblicati dalle riviste scientifiche. Proprio gli studi condotti in seguito alle controversie sulla sicurezza dei vaccini sono stati spesso

perché sono stati approvati degli emendamenti che non hanno migliorato il decreto-legge, ma lo hanno anzi peggiorato, aumentando la confusione. Ad esempio, all'articolo 1 è stato eliminato il vaccino per il *papilloma virus*, che rientrava

dipartimenti di prevenzione. È la ASL che, organizzandosi, deve dire chi deve fare la vaccinazione. Il personale della ASL è formato da anni ed è preposto a questo: si istituti di igiene. Va bene, invece, per praticità, applicare il discorso alle farmacie, ai sensi della legge n. 69 del 2010, ma nel decreto ministeriale dovrà essere ben dettagliato chi fa cosa e come e, soprattutto, occorre occuparsi dell'informatizzazione, in modo tale che i dati che i dati confluiscano nella rete nazionale delle vaccinazioni, che offre il dato delle coperture e anche il monitoraggio degli effetti avversi. Quel decreto ministeriale dovrà essere fatto con molto attenzione. È stato un altro errore tecnico

cosa non si è fatto? Non si è pensato a quello che sarebbe accaduto successivamente. Oggi, se una famiglia si rivolge alle ASL per fissare un appuntamento vaccinale, presso tante ASL ottiene

Altre richieste che abbiamo fatto al Governo sono state bocciate, come la seguente. Se avete imposto l'obbligatorietà, perché la richiesta della certificazione per poter iscrivere

Ma a parte il pagamento, che è un'assurdità, se c'è una obbligatorietà, e devo chiedere quella certificazione alla ASL o all'istituto ospedaliero che l'ha effettuata per portarla in una scuola, perché devo anche pagarla?

Le ASL trasmettono alle scuole i dati relativi ai ragazzi, con tutti i contenuti che avete deciso di chiedere. Era così difficile far funzionare il sistema senza creare altri oneri alle famiglie?

di una tale prescrizione. Voi dite che, siccome sono bambini non vaccinati, e tendenzialmente meno protetti, è bene che siano inseriti in una classe complessivamente protetta.

offriamo il destro perché questi bimbi, che si dice di voler proteggere, diventino ancora più vulnerabili.

proprio per proteggerla. E si tenga conto che un malato di HIV è estremamente pericoloso e può contagiare. Bene, se un ammalato di HIV ha la protezione, l'anonimato garantito per legge, non si capisce perché dobbiamo

la scuola, noi vorremmo che funzionasse. Conosciamo tutte le difficoltà e, a parte i decreti sulla buona scuola, che non so se abbiano veramente migliorato la funzionalità e la

in esame. Dovranno informare le famiglie, chiedere e ottenere la documentazione, fare le liste, provvedere: probabilmente accantoneranno i problemi della funzionalità scolastica, della copertura degli insegnanti, delle ore dell'insegnamento perché troppo rigida è l'imposizione che gli si dà

rendendo consapevole la popolazione, otteniamo risultati migliori che si avvicinano agli *standard* ottimali richiesti dall'Organizzazione mondiale della sanità, senza frizioni, senza sanzioni, senza esclusioni né ghettizzazioni dei ragazzi che sono non infetti ma soltanto - forse - un pericolo perché non vaccinati. Avete creato panico, le famiglie sono preoccupatissime e anche quelle che avrebbero portato naturalmente i figli a vaccinarsi adesso sono restie.

la famiglia capisce che qualcosa non funziona. Dovete recuperare la fiducia, dovete rassicurare le famiglie. I vaccini - lo ripetiamo - sono una cosa buona, ma bisogna farlo capire e non imporlo con la mannaia e con i vostri metodi.

Signora Presidente, voglio partire da due notizie di qualche settimana fa che mi sembrano molto significative per il dibattito complesso che stiamo affrontando. La prima: l'Accademia nazionale dei Lincei ha pubblicato un documento che si esprime in modo unanime e scientificamente documentato a favore dell'obbligatorietà dei vaccini. La seconda: l'OMS ha dato un cartellino giallo all'Italia per il calo della copertura media nazionale delle vaccinazioni, scesa sotto la soglia di sicurezza raccomandata. Aggiungo una terza considerazione. Con il provvedimento in esame l'Italia sta facendo quello che in California è successo un paio di anni fa, quando è stato reintrodotto l'obbligo dei vaccini per poter andare a scuola dopo un'epidemia grave di morbillo, che mise in pericolo di vita bambini leucemici che, non potendosi vaccinare perché immunodepressi, contrassero la malattia o furono costretti a non andare a scuola perché i compagni non erano vaccinati. Dopo la California molti altri Stati hanno seguito la stessa strada, e stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, il Paese più liberale del mondo. In Italia nel 1999 venne meno la legge che prevedeva la somministrazione di vaccini obbligatori ai bambini in età scolare. All'epoca era stato fatto un ragionamento: ormai tutti si vaccinano e quelli che non lo fanno sono pochissimi, dunque non creano problemi. Ma così purtroppo non è stato, e ora il Governo ha deciso di far di nuovo indossare la «cintura di sicurezza» chiamata vaccino, allacciandola anche ai bambini che hanno un tumore. E questa, io credo, sia una giusta decisione. Non ritengo uno scandalo, insomma, né un passo indietro dal punto di vista culturale, sanitario e sociale, che per iscrivere i propri figli a scuola torni ad essere necessario presentare il documento che attesta che il calendario vaccinale è stato rispettato. L'abbassamento della soglia di copertura in questi anni ha infatti favorito un aumento generalizzato dei casi di malattie infettive; basti pensare agli ultimi contagi da morbillo, che sono quintuplicati rispetto all'anno scorso. Le patologie sono arrivate a colpire fasce di età variegate, spesso diverse da quelle classiche, e quadri clinici più gravi, con maggiore ricorso all'ospedalizzazione e con conseguente aumento dei costi sanitari e sociali. Con questa premessa è chiaro che io sono d'accordo con la linea scelta dal Governo di tornare alle vaccinazioni obbligatorie, anche se era forse preferibile non intervenire attraverso un decreto-legge.

è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano si trasformino nel prossimo futuro in vere emergenze sanitarie. dunque, alla dichiarazione del Presidente del Consiglio, non c'è al momento una situazione di emergenza nazionale e pertanto non dovrebbero sussistere i presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Se, però, per effetto della campagna di vaccinazioni, può essere salvata anche una sola vita umana o si può prevenire il manifestarsi di inconvenienti particolarmente nocivi alla salute, allora può essere giustificata anche l'adozione del decreto-legge. C'è però un'incongruenza che mi preme segnalare: non è chiara infatti la *ratio* del diverso regime stabilito per asili nido e materne, da un lato, e scuola dell'obbligo, dall'altro: condizione dell'iscrizione l'avvenuta somministrazione del vaccino nel primo caso, obbligatoria anche nel secondo caso, ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata effettuazione. Due osservazioni al riguardo; la prima è che tanto l'interesse all'istruzione, quanto quello alla salute, si appuntano in capo ai singoli come pure alla collettività. Non si capisce se e come essi siano stati bilanciati in questo decreto-legge. Se c'è infatti il rischio di contagio di malattie diffusive, anche per la scuola dell'obbligo dovrebbe essere necessaria la vaccinazione quale condizione dell'iscrizione. Se, al contrario, il rischio non c'è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di essere salvaguardato il diritto all'istruzione fin dalla scuola materna. Sarebbe stata poi molto complessa la questione dell'eventuale sospensione della potestà genitoriale, che in Commissione è stato proposto giustamente di depennare. La giurisprudenza costituzionale al riguardo ci ha infatti ripetutamente insegnato che ogni automatismo legislativo, quale quello che al ricorrere di alcune circostanze di particolare gravità porti alla perdita della potestà genitoriale, si scontra col preminente interesse del minore, che va sempre e comunque salvaguardato. C'è un ultimo rilievo, rivolto nelle passate settimane al decreto-legge, che merita di essere approfondito. Si aumenta il numero di vaccini obbligatori da quattro secondo il Codacons, la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini ad una dose massiccia di vaccini senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale con conseguente e possibile incremento delle reazioni avverse. Una situazione che potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge venisse sottoposto al sindacato della Corte costituzionale. Tutti dubbi legittimi, visto che stiamo trattando una questione particolarmente complessa, che tocca i rapporti tra scienza, etica e diritto.

Per questo, auspicando che il Governo non ponga la questione di fiducia per lasciare aperta la porta a ulteriori miglioramenti emendativi, annuncio già da ora il mio voto favorevole al provvedimento, anche nel caso in cui il mio Gruppo decida in modo diverso. *(Applausi del

vari capitoli e varie indicazioni per renderlo attuabile e fare in modo che la percentuale dei bambini vaccinati si alzi nell'interesse più generale del termine. In linea generale, personalmente non sono mai favorevole all'obbligatorietà per quanto riguarda le decisioni sulla famiglia o la salute del proprio bambino. Vorrei ricordare che uno degli aspetti che verranno discussi successivamente è il consenso informato. Per cui, la nostra opinione è che dovremmo fare un'azione di convincimento nei confronti dei cittadini e delle famiglie per fare in modo che ai bambini venga assicurata una vaccinazione che li ponga al riparo dalle malattie infettive non solo per se stessi, ma anche per altri e, cioè, per garantire la salute in senso più generale. Al contrario, in questo decreto-legge, su alcune questioni, il comportamento non è proprio così. che da un punto di vista scientifico viene detto che, spesso e volentieri, la trasmissione delle malattie avviene anche e non soltanto tra bambini e bambini, ma anche tra adulti e bambini, noi riteniamo che debba essere tenuto in considerazione il fatto

bambini. Ciò non è stato fatto; si era pensato a campagne di informazione sul *fertility day* e abbiamo visto come è andata a finire. C'è anche un problema di scelte di priorità

Abbiamo un Ministro della salute che ci dice che c'è un'emergenza per cui bisogna intervenire con decreto-legge perché ci sono delle epidemie e c'è il Presidente del Consiglio che, al contrario, sostiene che non ci sono emergenze, non ci sono epidemie e che l'eventuale epidemia

soprattutto di esame degli emendamenti si possa trovare una via d'uscita a tutto questo; a condizione però che non ci venga proposto di ritirare gli emendamenti per trasformarli in raccomandazioni, perché sappiamo benissimo che fine fanno gli ordini del giorno e le raccomandazioni. C'è quindi apertura al dialogo, ma

Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, il decreto-legge ora in discussione è motivo di grande perplessità per molti esperti, professionisti e per molte famiglie ed ha aperto un dibattito molto delicato che avremmo forse dovuto evitare. Anche io credo che in premessa sia opportuna una precisazione: la mia posizione è a favore dei vaccini sicuri ed efficaci. La validità delle vaccinazioni come mezzo di prevenzione delle malattie infettive è universalmente riconosciuta (salvo pochissimi casi che si condannano) dalla comunità scientifica e dalla cittadinanza informata. Ogni obiezione di principio sarebbe inutile e fuori luogo; non vi sono dubbi che le vaccinazioni hanno contribuito al progresso della medicina e che continuano a contribuire alla riduzione della morbilità e della mortalità, soprattutto in Paesi ad alta prevalenza di malattie trasmissibili. Proprio per questo ritengo che ogni decisione su una materia tanto importante per la salute del singolo individuo e della collettività debba essere presa tenendo conto delle più aggiornate e robuste evidenze scientifiche disponibili e del contesto in cui si calano. Questo è quanto affermato anche dalla Organizzazione mondiale della sanità. A fronte di questa premessa non si può peraltro non rilevare che nell'attuale dibattito sulle vaccinazioni sembrano prevalere fattori culturali, politici ed economici che rischiano di avere più peso delle evidenze scientifiche. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un susseguirsi di dichiarazioni anche contrastanti, ancorché fatte dalla stessa persona, e prive di robuste motivazioni, provenienti da persone che per il loro ruolo dovrebbero sentirsi tenute (soprattutto su un tema così delicato, ma in generale sempre) alla massima obiettività, evitando facili slogan e senza alimentare contrapposizioni radicali e divisioni del Paese. Proprio perché non si può rischiare di depotenziare il ruolo delle vaccinazioni sicure ed efficaci ritengo si debba evitare in ogni modo di adottare provvedimenti che possano aumentare il problema delle esitazioni vaccinali, che è noto a livello internazionale. Negli ultimi anni è stato studiato e denominato scetticismo vaccinale dall'Organizzazione mondiale della sanità, la quale ha affermato che per comprendere il fenomeno bisogna studiarne le cause, le cause, che sono da ricondurre a tre sostanziali fattori che si sommano: la mancanza di fiducia nelle vaccinazioni purtroppo c'è, non possiamo che prenderne atto anche se possiamo volerla contrastare; la difficoltà da parte di tanti giovani genitori a prendere una decisione impegnativa per il proprio figlio (che dobbiamo comprendere, perché fa parte dell'ansia di crescere un figlio);

Ora, possiamo pensare che queste cause indicate dall'Organizzazione mondiale della sanità con riferimento ai Paesi sviluppati siano alla base del calo delle coperture vaccinali anche nel nostro Paese? Credo proprio di sì e molti esperti lo dicono. Se è così, quali azioni lo Stato e le Regioni avrebbero potuto e possono adesso mettere in opera per contrastare questa tendenza? L'azione necessaria è lavorare per far recuperare la fiducia della cittadinanza nelle indicazioni provenienti dalle istituzioni sanitarie. La disinformazione, la scarsa fruibilità dei dati, l'utilizzo di termini troppo complicati, la paura di eventuali effetti collaterali sono tutti fattori che in qualche modo andrebbero aggrediti da chi ha la responsabilità della tutela della salute. Ascoltare i genitori, produrre informazioni facilmente comprensibili, oggettivare sempre benefici e rischi delle vaccinazioni: questi sono gli ingredienti che non vanno improvvisati e non vanno dimenticati. Essi sono costitutivi di quel rapporto di fiducia che sta alla base, fin dalla nascita del bambino, del rapporto fra medico, operatori sanitari e cittadini; ed è solo dentro questa relazione che è possibile dialogare serenamente e favorire una decisione consapevole e responsabile, delicata proprio perché relativa non solo al proprio figlio, ma anche ai suoi rapporti con il resto della collettività. Sarebbe anche necessario riconoscere che il tempo dedicato a questa relazione è vero e proprio tempo di cura. Questo è importante, ma l'abbiamo troppo spesso dimenticato; gli operatori alla fine non dedicano più tempo a questi aspetti. Lo scetticismo vaccinale però è legato anche ad altri fattori, che non dovrebbero essere trascurati, né tanto meno rimossi, anche quando purtroppo ci feriscono, perché rischiano di intaccare delle convinzioni profonde che abbiamo e che vorremmo mantenere tali. Fatti come la frettolosa e colpevole pubblicazione, in una prestigiosissima rivista scientifica internazionale, di un articolo sui danni da vaccini vaccini (poi rivelatosi privo di qualunque fondamento e quindi ritirato dalla stessa rivista, ma ormai aveva prodotto effetti devastanti sul comportamento delle persone) producono effetti enormi, sui quali la comunità scientifica per prima, anziché rivendicare soltanto la correttezza sempre e comunque della scienza, dovrebbe interrogarsi e si sta interrogando. Ma forse lo dovrebbe fare con ancora maggiore forza. poi i casi di allarmi di epidemie e anche di pandemie, poi rivelatisi infondati, così come i casi accertati corruzione oggetto di condanna in via definitiva, che purtroppo hanno riguardato anche il nostro Paese. Questi temi non fanno che aumentare i dubbi e i timori delle persone e mettono a dura prova la credibilità delle istituzioni, di tutte le istituzioni: quelle politiche, quelle scientifiche e, soprattutto, quelle sanitarie. Per non parlare poi dell'uso di Internet, che spesso viene considerato il principale colpevole, ma che in realtà non è l'unico. Ebbene, da molti anni tutti, a partire dal Governo, avrebbero dovuto mettere in atto azioni di contrasto di questi fenomeni, perché li conosciamo da molti anni è sappiamo che bisogna tentare di contrastarli. Azioni ben disegnate avrebbero potuto forse contenere, magari soltanto in parte, la crescita delle esitazioni, ma certamente non sarebbero state inutili. E invece, a quanto ci risulta, le grandi ristrettezze cui sono state sottoposte le aziende sanitarie e le condizioni di accesso ai servizi vaccinali, che sono in molte parti inaccettabili (lo sappiamo bene, dalla Lombardia alla Sardegna ci vogliono mesi e mesi per prenotare la vaccinazione di un bambino, le vaccinazioni sono in molti territori sottoposte a *ticket* e così via), sono tutti fenomeni che non aiutano i genitori a prendere le decisioni in modo adeguato. Non posso non ricordare che la lenta riduzione delle coperture vaccinali ha avuto inizio intorno al 2013. In questi quattro anni forse qualcosa di più avrebbe dovuto essere fatto e avrebbe anche potuto essere fatto, in primo luogo a partire dal Governo. non mi si venga a dire, come spesso mi è stato risposto, che questo è compito delle Regioni: lo Stato ha il compito di monitorare l'erogazione dei livelli essenziali e di intervenire in caso di inadempienza delle Regioni, e i vaccini sono parte dei livelli essenziali. Da tempo anche in Commissione sanità, all'unanimità delle componenti partitiche, abbiamo denunciato le debolezze con le quali il livello centrale svolge la funzione di monitoraggio e di intervento in caso di inadempienze rispetto ai livelli essenziali. veniamo al merito del decreto-legge. Il primo aspetto riguarda la coerenza rispetto alla programmazione sanitaria vigente, in particolare il piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, che è stato approvato a gennaio del corrente anno e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio scorso. Tale piano è impostato su una visione che fa «dell'educazione sanitaria, della responsabilizzazione e dell'*empowerment* dei cittadini» il fulcro di tutte le azioni da intraprendere al fine di tutelare la salute della popolazione, anche attraverso lo strumento delle vaccinazioni. Non emerge in quel documento una presa di posizione chiara e generalizzata verso l'obbligatorietà dei vaccini come unico strumento da adottare in caso di preoccupazione, mentre questo lo si legge nel decreto-legge; eppure, i dati di copertura vaccinale erano noti da tempo e non erano molto dissimili da quelli di oggi. Qual è la ragione di un tale cambiamento di rotta? Evidentemente gli estensori dei due documenti non si sono coordinati tra loro; non ci sono altre spiegazioni ragionevoli.

ulteriore rispetto a un panorama già molto differenziato a livello regionale e che certamente non ammette che la risposta sia che tutte e tre le soluzioni hanno forti fondamenti scientifici: ne può valere solo una delle tre; oppure ci sono degli elementi di distinguo - che riteniamo ci siano - che dovrebbe essere esplicitati. Una seconda questione riguarda l'effettiva necessità di un provvedimento urgente su dodici vaccini. Anch'io ho considerato la necessità di procedere nel merito nei confronti del decreto-legge ma i dati disponibili per il nostro Paese, che purtroppo non sono chiari e facilmente accessibili, segnalano un calo delle coperture vaccinali al di sotto della soglia raccomandata dall'OMS del 95

Tale livello critico costituisce motivo di preoccupazione soltanto per il morbillo.

affrontando le altre situazioni di preoccupazione debole con gli altri strumenti di promozione attiva di un'adesione volontaria e consapevole? II caos del morbillo mette in evidenza un altro problema: la necessità che l'obbligo, se siamo convinti ci sia un'emergenza, sia esteso a tutti gli operatori della sanità e forse anche ad età successive a quelle della scuola dell'obbligo. delle persone colpite da morbillo è di ventisette anni e sappiamo che ci sono casi di morbillo che transitano attraverso gli operatori sanitari. Qui lo so qual è la risposta: è un problema di copertura.

oppure non c'è un problema di emergenza per il morbillo (e allora usiamo la stessa azione nei confronti dei bambini e - almeno - degli operatori della sanità).

anti-meningococco B e C, che poi fortunatamente, in occasione del dibattito in Commissione, sono stati trasformati in vaccini solo raccomandati? Perché non si è lavorato di più - qualcosa è stato fatto e ringrazio - per semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini? Perché il decreto-legge non contiene nulla sulla farmacovigilanza e sugli archivi vaccinali è stata introdotta in Commissione)? Come si fa a pensare che ci sia sufficiente rigore scientifico e attenzione in un decreto-legge che non guarda alle applicazioni? Perché, ancora, non consentire la rifinalizzazione delle risorse che, con la legge di bilancio approvata nel dicembre scorso, vincolato all'acquisto dei vaccini all'intera realizzazione del programma vaccinale? Che senso ha soprattutto nei primissimi anni, o almeno nel primo anno di applicazione della norma, acquistare vaccini, quando sappiamo che ci sono strutture non in grado di somministrarli per carenza di personale

per l'Istituto di sanità pubblica diretto dal professor Gualtiero Ricciardi, che attualmente è in aspettativa perché Presidente dell'Istituto superiore di sanità. Tale Istituto e, in in prima persona, il professor Ricciardi sono stati i superesperti che hanno consigliato il Ministro in tutte le questioni relative alle vaccinazioni. Il finanziamento di questa cattedra è a carico di privati, la Merck Sharp & Dohme, che è l'azienda *leader* nella lotta contro le malattie prevenibili con vaccinazioni e nella produzione dei vaccini. Siamo ancora in attesa di risposte di merito. Mi permetto di offrire brevemente qualche ultima riflessione. Per quanto capisco, il tema di cui ci stiamo occupando sembra attenere più a questioni di concorrenza politica ed elettorale elettorale e nella ricerca del consenso e dei finanziamenti, nonché di compiacenza nei confronti di alcuni poteri (da quelli economici a quelli politici) e di aspirazione a specifici benefici, remunerazione per prestazioni aggiuntive. È iniziata la corsa, tutti vogliono approfittare dei programmi di vaccinazione per avere delle risorse. Vi sono inoltre risorse per cattedre universitarie e nuovi ruoli per alcuni professionisti, a partire dalle farmacie private. Gli aspetti inerenti alla protezione contro le malattie infettive prevenibili sembrano essere - mi auguro di sbagliare - il mezzo, anziché il fine. la mancata risposta su questi importanti aspetti lascia purtroppo aperti tutti i quesiti sul perché dell'accanimento inflessibile da parte del Governo nella difesa dei pilastri fondamentali dell'impianto del decreto-legge. Noi non sottovalutiamo l'importanza delle vaccinazioni. Nessuno vuole istituzioni indifferenti alle epidemie, ma la gestione dei rischi richiede capacità di analisi, di intervento, indipendenza e robusta capire le esitazioni delle tante giovani mamme che chiedono trasparenza. Ancora un ultimo aspetto. Ringrazio la Commissione, come ho già detto, per l'impegno e il lavoro svolto e per i miglioramenti introdotti. Mi resta l'amarezza - lo devo dire apertamente - per la disattenzione con la quale il Governo

a favore degli interventi dei medici di medicina generale e dei pediatri e non a favore degli operatori e dei dipendenti della sanità che lavorano nei centri vaccinali. significa che non ha a cuore l'applicazione di questo provvedimento e forse neanche la mortificazione di cui stanno soffrendo molti operatori della sanità.

Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, Aula vuota e piazze piene. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che l'Assemblea, nei momenti di discussione generale, è a ranghi ridotti; ma mi permetto di osservare che in questa occasione avrei preferito che vi fosse una presenza più numerosa, per sviluppare quel senso di auspicata responsabilità che deve accompagnare la decisione e il voto su un provvedimento particolarmente complesso. Complesso al punto tale che mi sono chiesto più volte se giusto che provvedimenti ad alto livello di complessità sotto il profilo tecnico e scientifico, dove i profili di natura scientifica prevalgono sulle valutazioni di tipo politico, politico, arrivino in Aula e non si proceda invece con provvedimenti differenti, con leggi di delega, ben palettate, ma naturalmente consegnate a una decisione sottratta alle condizioni di emotività.

Eppure accade questo quando la forza della pancia riesce a condizionare e a orientare il voto su provvedimenti delicatissimi come questo non solo non si rende un buon servizio alla qualità del nostro sistema sanitario nazionale e alla tutela della salute, ma non si rende un buon servizio neanche alla democrazia. Il tema è delicato e complesso e quando si parla di farmaco accade quasi sempre, quasi sempre, perché esso occupa una posizione trasversale, con le sue numerose implicazioni rispetto ai vari risvolti, che sono senz'altro quelli più percepiti, di natura tecnicoscientifica, connessi con il pilastro a cui i ragionamenti devono ispirarsi, ossia quello della scienza; ma vi sono anche altre implicazioni, di natura culturale, sociale, economica, etica, forse addirittura antropologica.

sue antinomie: indicazioni e controindicazioni, benefici e rischi, promessa di salute ed effetti collaterali, uso ed abuso, in riferimento alla disobbedienza. Quindi ci sono anche contraddizioni e paradossi: ne abbiamo visti ed ascoltati, nei giorni e nei mesi scorsi e lo facciamo ancora oggi in quest'Aula.

le piazze si sono mobilitate, paradossalmente, per consentire l'accesso a cure con presunti farmaci e per stimolare il legislatore ad eliminare divieti, vincoli e preclusioni rispetto a metodiche terapeutiche frutto di una ciarlataneria, che impera. In passato abbiamo visto le piazze che sollecitavano il "palazzo" a consentire l'uso del siero di Bonifacio, del metodo Stamina di Vannoni, della cura Di Bella, senza che vi fosse una fondatezza scientifica in merito a questi metodi presuntamente terapeutici. rivoluzioni di piazza con crociate antiscientifiche, con una incitazione all'uso di sostanze prive di efficacia riconosciuta e forse dannose. per ultimo e non da ultimo, il caso del "Vidatox", il veleno di scorpione, su cui abbiamo svolto un'indagine conoscitiva. Voglio ricordare l'indagine conoscitiva sul metodo Stamina, che ha portato a conclusioni inequivocabili, che hanno trovato riscontro anche nell'arresto del sostenitore di questo tipo di metodica. Il paradosso è che da una a presunte terapie farmacologiche prive di fondamento scientifico, mentre oggi ci sforziamo in tutti i modi di diffondere una perversa, preoccupante e dannosa cultura di disinformazione sul valore e sul significato della vaccinazione. Non sento una parola, da parte del popolo "No vax" sui 68 morti che ogni giorno vengono consegnati alle statistiche epidemiologiche e che periscono sotto i colpi profondi delle antibiotico-resistenze. Sto parlando di 68 morti al giorno, secondo i dati confortati dalle massime autorità di settore in ambito europeo. Sebbene l'Italia detenga il consumo più elevato di antibiotici, non c'è un intervento

accompagna la storia dell'uomo. Le ragioni, un po' religiose e un po' ideologiche del "no" riassorbono e riassumono le stesse ragioni per cui, alla fine dell'Ottocento, si tentò di invalidare la ricerca scientifica e le grandiose intuizioni di Edward Jenner, che aprì l'era delle vaccinazioni.

Diffondiamo, attraverso la cultura del sospetto e delle insinuazioni, uno scetticismo dannosissimo che ci allontana dal traguardo. Mi permetterei di dire anche che quella valanga di insinuazioni, sulle robuste spalle di autorevoli ricercatori e persone delle istituzioni, sono un'offesa che va oltre il riferimento alle singole persone. I vaccini sono il più efficace intervento medico dopo la potabilizzazione dell'acqua: lo dice l'OMS. I vaccini costituiscono ancora oggi la migliore misura di prevenzione, perché il rapporto rischio-beneficio è assai positivo e con un valore non solo sanitario, ma mi permetto di dire anche etico, perché la cultura della vaccinazione è cultura della solidarietà:

aspetti epidemiologici. Certamente possono esserci eventi avversi, ma c'è un sistema di farmacovigilanza che nel nostro Paese funziona e si evolve anche attraverso recenti recepimenti di normative comunitarie che hanno previsto un sistema proattivo

della speculazione politica per pareggiare i conti. Credo infatti che un simile ragionamento - parlo da forza di opposizione - non vada nella direzione di sostenere le ragioni della tutela della salute collettiva, in un Paese civile che oggi viene messo in coda nelle classifiche internazionali sui livelli di copertura vaccinale. Certamente esistono delle criticità, ad iniziare dallo strumento utilizzato che è il decreto.

avrebbero potuto lasciare spazio a una riflessione e a un confronto maturo, qualificato, responsabile e approfondito per superare alcune criticità che restano. Il decreto rappresenta infatti uno strumento imperativo, in termini di metodo, ma imperativi sono anche i contenuti. Avrei preferito, rispetto all'introduzione dell'obbligo, che pure per alcuni versi è necessario, avesse prevalso la promozione di una forte campagna di educazione, informazione e sensibilizzazione, che rappresentano parole d'ordine per recuperare quel livello di distensione e pacificazione che invece non trova riscontro in un Paese che si sta inopinatamente dividendo tra *pro* e contro i vaccini.

il vaccino monocomponente. Perché è necessario fare la trivalente e non si ricorre all'uso del vaccino monocomponente? Impegniamoci a capire perché non si trova in commercio il monocomponente. Anche le fasce *target* vanno aumentate: è stato detto che l'età mediana per il morbillo è l'obbligo vaccinale per gli operatori; la copertura vaccinale per gli immigrati; l'accesso ai servizi vaccinali in termini di idoneità degli ambienti e tempi di accesso. L'emendamento sulla possibilità delle vaccinazioni in farmacia è figlio di una grave carenza sotto il profilo strutturale, tecnico, organizzativo, degli organici e di ambienti fatiscenti. L'afflittività delle sanzioni è uno degli aspetti ai quali noi attendiamo che il Governo destini un'attenzione maggiore in un recuperato rapporto rapporto di responsabilità reciproca, evitando che si consolidi quello strappo interno al Paese che sta determinando un danno finanche alla nostra democrazia su un tema

della medicina della evidenza e del rigore scientifico. Signor Presidente, cari colleghi, la legge in discussione è importante, una delle più importanti leggi di sanità pubblica della legislatura, quella che più di tante altre migliorerà le prospettive di salute dei cittadini italiani. Al ministro Lorenzin, al Governo nel suo insieme, alle Commissioni e alla relatrice va il mio riconoscimento per aver saputo trattare con responsabilità e lungimiranza le politiche di salute pubblica, senza temere critiche immotivate e guardando al benessere dei cittadini di domani. Anche io, come tutti voi, ho ricevuto messaggi di ogni tono e contenuto, ho letto notizie non sostanziate, che alimentano paure umanamente comprensibili ma scientificamente insensate. Hanno ragione la senatrice Maturani e il senatore Buemi nel ricordare che questi sono comportamenti che nascono, probabilmente, anche dalla percezione che le malattie che falcidiavano le generazioni che ci hanno preceduto fortunatamente non sono più intorno a noi. Non abbiamo più davanti agli occhi la tragica testimonianza di persone colpite da poliomelite o da vaiolo, ma *virus* e batteri non sono affatto spariti. Molti infettano l'uomo per rigenerarsi. Li abbiamo intorno, li possiamo e li dobbiamo tenere sotto controllo, senza abbassare la guardia, dando il nostro contributo anche nell'informare, sapendo che informare su questioni di scienza può non essere facile. facile. Il nostro cervello, infatti, funziona in modo un po' strano e questo ce lo spiega chi si occupa di psicologia cognitiva e di neuroscienza cognitiva. Il nostro cervello ha forti pregiudizi, retaggio della sua storia evolutiva lunga decine di migliaia di anni, quando doveva pensare alla sua individuale sopravvivenza e a reagire alle emergenze del subito mentre esplorava la savana del pleistocene. Ebbene, gli storici della medicina e gli psicologi cognitivi ci spiegano che il nostro cervello è uscito dalle caverne solo diecimila anni fa questa è una citazione dai loro testi - quando stava in altri contesti e fa fatica, oggi, con informazioni scientifiche che parlano di prevenzione quindi, di anni che verranno, quando prima gli anni non esistevano), di probabilità, di statistica, di rapporto rischi-benefici e di precauzione. Fa proprio fatica: è come se il nostro cervello fosse proprio inadatto a ragionare su questi temi. Quindi, è vero che informare è importante, ma informare non basta. Vi sono già studi, proprio su famiglie che non vogliono vaccinare i propri figli, che dimostrano che una informazione correttiva è utile con una parte dei dubbiosi ma addirittura controproducente con i più scettici. Questi studi ci dicono, e dovrebbero davvero allenarci sulle politiche, su come informare, che è sbagliato correggere i falsi miti o rimuovere gli errori di giudizio così radicati nel nostro cervello evolutivo, perché così si stimola quello che è noto come *backfire effect* cioè l'effetto del ritorno di fiamma o il *bias* di conferma che rafforza il rifiuto. Così forse ci spieghiamo le radicalizzazioni delle posizioni. Ecco, quindi, che non si devono rimuovere le convinzioni sbagliate, ad esempio che i vaccini causano l'autismo, ma si deve dare una nuova informazione e dire, cioè, cosa succede a un bambino colpito colpito dal virus della parotite o della rosolia. Questa modalità informativa si è rivelata efficace in una parte degli scettici. Quindi, non abbassare la guardia significa anche sviluppare modi per informare su tematiche di salute pubblica e chiarire le questioni più dibattute. Lo farò anch'io citandone alcune, con il supporto della logica, delle prove e della letteratura scientifica più recente. La prima questione riguarda la difesa, da più parti richiamata, della libertà individuale; ma invocarla in questo contesto è come sostenere che ognuno deve essere libero di togliere i freni alla propria auto perché sospetta che siano stati disegnati male, sostenendo di poterne fare a meno schivando ogni ostacolo o frenando con i piedi. Non si può invocare la libertà di mettere a rischio la vita altrui. La seconda questione riguarda, invece, la nostra responsabilità sociale e collettiva di cittadini: responsabilità che deriva dalla cosiddetta immunità di gregge, più volte richiamata, con la quale la comunità si autoprotegge dall'insorgenza della malattia perché la circolazione dell'agente patogeno diventa impossibile. Questa soglia di sicurezza raccomandata dall'OMS varia a seconda del tipo di malattia ed è pari al 95 per cento, per esempio, nel caso del morbillo. Si è già sottolineato in questa Assemblea che rifiutare le vaccinazioni, facendo abbassare questa soglia, significa esporre a rischi letali i propri figli e quelli altrui, bambini in età prevaccinale o bambini e adulti con un sistema immunitario compromesso a causa di malattie autoimmuni o tumori. Rifiutare Rifiutare le vaccinazioni significa anche lasciare il patogeno libero di infettare le cellule dell'organismo, quindi di modificarsi per dare origine a ceppi più virulenti e mutati per i quali i vaccini attuali potrebbero non funzionare. Quindi, un individuo non vaccinato può funzionare da veicolo per la creazione di ceppi resistenti agli attuali vaccini. Il terzo punto riguarda l'affermazione per cui l'Italia sarebbe l'unico Paese in Europa a ricorrere all'obbligo per un numero così elevato di vaccini. Eppure, quando si sono presentati dei cali delle vaccinazioni, i diversi Paesi hanno reagito e hanno preso sempre provvedimenti. La Germania ha introdotto sanzioni economiche per i genitori che non segnalano alle autorità il loro rifiuto di vaccinare i figli al momento dell'iscrizione al nido. In Francia sono stati resi di nuovo effettivi alcuni provvedimenti legali e due genitori, che senza motivata ragione - se non le personali percezioni si sono opposti alla vaccinazione per i loro figli, sono stati sanzionati. Un mese fa, sempre in Francia, si è aperto un dibattito per rendere obbligatorie 11 vaccinazioni pediatriche, rispetto alle attuali tre. Non c'è dubbio che l'obbligo deciso per decreto-legge sia un'emergenza, una scorciatoia per riportare la copertura vicina alla soglia di sicurezza; ma è la decisione più veloce ed economica per raggiungere i tassi di copertura suggeriti dall'OMS. Al senatore Divina, che mi sembra sostenere che l'obbligo non sia necessario perché non ci sono epidemie in atto, mi viene da rispondere: meno male. Con questo provvedimento ci si affida alla medicina proprio per prevenire un tale e sciagurato epilogo al Paese. Il quarto passaggio riguarda la presunta pericolosità dei vaccini. Negli ultimi vent'anni non ci sono state morti scientificamente correlabili ai vaccini. Quante, invece, le persone decedute a causa di malattie infettive considerate scomparse! Nel XX secolo, quando i vaccini non esistevano, quasi 1,7 miliardi di persone sono morte per malattie infettive e la nostra aspettativa di vita è passata dai agli ottantacinque odierni, grazie alla sconfitta di tante malattie dovute anche ai vaccini, oltre che a una migliore igiene e all'uso di antibiotici. Nel mondo occidentale le vaccinazioni di massa hanno evitato la morte di 500 milioni di persone e pensate che nell'attuale decennio 2011-2020 permetteranno di evitare la morte di 25 milioni di persone. Come tutti i farmaci anche i vaccini possono causare reazioni avverse. Ci possono essere alcune, rarissime, reazioni gravi, comunque trattabili, come anafilassi, dolori articolari, edemi, per le quali è previsto il ricovero temporaneo; parliamo però di meno di un caso su un milione e, nel complesso, l'incidenza delle reazioni avverse è inferiore a quella dei più banali farmaci in commercio. esempio, causa un numero di reazioni avverse 1.500 volte maggiore dei vaccini. Sempre circa la pericolosità, ricordo in quest'Aula la nota frode scientifica del chirurgo britannico Wakefield. Egli sosteneva che a seguito della vaccinazione trivalente, alcuni bambini avessero contratto l'autismo. Ma due eventi in sequenza non sono necessariamente collegati. Quella di Wakefield fu una frode inventata per interessi economici, scoperta da un giornalista e poi smascherata da studi scientifici che hanno sempre smentito le correlazioni tra vaccinazioni e autismo, una malattia difficile che oggi sappiamo avere tratti di natura genetica, con i primi segni in epoca fetale e quindi prevaccinazione. Pensate però che quel tragico inganno ci offre un esempio di cosa succede quando si è in presenza di un calo delle vaccinazioni; ci fu l'esplosione di un'epidemia nel Regno Unito nel 2012, con quasi 10.000 casi di parotite, la morte di 15 bambini, un'epidemia di morbillo, ospedalizzazioni e casi gravi. È la prova drammatica di come la pseudoscienza possa diventare un pericolo concreto. Come quinto punto, vorrei dare una risposta all'interrogativo relativo al numero di vaccini resi obbligatori, da molti ritenuto eccessivo per un bambino. Molti dati indicano che non c'è da preoccuparsi. Un antigene è un piccolissimo pezzo di microorganismo. È, in altre parole, una singola sostanza dotata di proprietà immunogeniche, in grado cioè di stimolare il nostro sistema immunitario. Con un graffio o una puntura di zanzara un bambino entra in contatto istantaneamente con migliaia e migliaia di antigeni. Fino a pochi anni fa i pochi vaccini di cui disponevamo contenevano 3.000 antigeni. Pensate che oggi, con più vaccini, siamo scesi a meno di 100 stimolazioni e, quindi, a meno di 100 antigeni. L'ultimo punto riguarda i presunti interessi delle case farmaceutiche ad alimentare il mercato dei vaccini. Un documento del 2015 dell'Agenzia del farmaco sui costi dei vaccini per il nostro Sistema sanitario nazionale sottolinea come in quell'anno la spesa nazionale per i vaccini fosse stata l'l,4 per cento della spesa totale del sistema sanitario per i farmaci e la situazione non è diversa in Europa. La preoccupazione è anzi che oggi solo 5 case farmaceutiche producono la maggior parte dei vaccini,

Il dibattito sui vaccini ci impone infine una riflessione sul nostro sistema di giustizia. È probabile che l'applicazione della legge che ci accingiamo a votare investirà presto i tribunali italiani. Il caso Di Bella prima e Stamina poi ci hanno insegnato che il nostro sistema di giustizia si presta alla possibilità di ignorare le direttive delle autorità sanitarie. Per questo nel 2015, la Commissione Sanità del Senato, al termine dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Stamina, aveva proposto all'unanimità di prevedere il coinvolgimento dell'autorità sanitaria competente nei giudizi che riguardano la sperimentazione di farmaci. Oggi abbiamo l'opportunità, con questa legge, di renderlo effettivo. Grazie al sostegno del Gruppo delle Autonomie e di singoli colleghi appartenenti alle diverse forze politiche del Governo, è stato approvato l'emendamento che prevede il coinvolgimento nel processo dell'Agenzia italiana del farmaco nel caso di controversie relative ai farmaci, siano essi vaccini o farmaci oggetto di sperimentazione. Si tratta di una norma che vorrei dedicare alla memoria del professor Paolo Bianco dell'Università La Sapienza e del Generale dei NAS Cosimo Piccinno. Uomini delle nostre istituzioni, di cui abbiamo conosciuto le competenze e l'inesauribile determinazione nell'aiutare il Paese e la giustizia nel far emergere la verità nella cosiddetta vicenda Stamina. Nel ricordo della loro passione civile, e ferma restando la piena autonomia del magistrato, con la norma «Bianco-Piccinno» si prevede la presenza obbligatoria nei processi della massima autorità in materia, che dovrebbe limitare il rischio che si ripetano giudizi scientificamente infondati, come successe in troppi processi proprio su Stamina. In altri termini, questa norma cerca di prevenire scelte improprie su quel che ci è più caro: la salute. Cari colleghi, approviamo questo provvedimento, ma non consideriamo un traguardo l'aver sancito un obbligo. Il vero traguardo l'avremo raggiunto quando, imparando a informare i cittadini su questo tema, ne avremo fugato i timori e riconquistato la fiducia. Quest'opera, prima ancora della comunità politica, impegna tutta la comunità medica e scientifica, così come gli umanisti, della cui fondamentale funzione divulgativa e partecipativa alla vita democratica del Paese non mi stancherò mai di affermare la necessità. La scienza, ricordiamolo, lavora per il benessere di tutti, ma perché essa sia condivisa e accettata

Signor Presidente, egregi colleghi, se dovessimo farci guidare nell'esprimere il nostro voto dalla quantità di *mail* contrarie ai vaccini e alla loro obbligatorietà che abbiamo ricevuto in questi giorni, non avremmo dubbi e voteremmo no. Ma sono effettivamente l'espressione del sentire comune del nostro Paese o piuttosto il frutto del dilagare negli ultimi anni di un'informazione priva di supporto scientifico, portata avanti da soggetti privi di ruolo e di competenze all'interno del Sistema sanitario nazionale? Non ci troviamo forse di fronte alla classica situazione di una maggioranza silenziosa che subisce mentre vengono amplificati dal *web* messaggi allarmanti e preoccupanti sull'utilizzo dei vaccini e vengono diffuse notizie prive di fondamenti ritengo opportuno richiamare le prese di posizione di alcuni organismi autorevoli e con competenze specifiche. Recentemente, l'Associazione culturale dei medici pediatri ha sollevato il problema dell'esistenza in Italia di un sistema vaccinale non uniforme tra le varie Regioni con diversità di piccola entità in alcuni casi, ma anche in misura molto rilevante in altri, chiedendo l'istituzione di un sistema vaccinale unico. L'Organizzazione mondiale sella sanità (OMS), a proposito di questo decreto, di fronte al calo della copertura vaccinale in Italia, ha manifestato la propria preoccupazione per l'espansione dei casi di morbillo e di altre malattie prevenibili, garantendo il proprio supporto tecnico per migliorare la copertura e raggiungere il controllo delle malattie che minacciano di ripresentarsi a livello epidemico. L'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità hanno recentemente lanciato l'allarme per la forte riduzione delle coperture vaccinali nella popolazione; una così forte riduzione equivale a interrompere il processo di prevenzione avviato con la copertura vaccinale di massa, con la conseguenza gravissima del ripresentarsi di malattie eliminate da anni. Richiamo poi le recenti decisioni dell'ordine dei medici italiani, che hanno portato alla radiazione dall'ordine di alcuni responsabili di prese di posizione contrarie alle vaccinazioni. Ma quanti sono i casi esaminati? Tre su oltre 300.000 medici. Eppure per tre medici è stata messa in moto una sorprendente grancassa mediatica. Sottolineo anche un elemento che rischia di passare inosservato: negli ultimi anni sono notevolmente aumentati gli spostamenti e le migrazioni con conseguente aumento di contatti tra persone provenienti da Paesi diversi e connesso rischio di trasmissione di agenti patogeni di malattie trasmissibili. Inoltre, in alcune zone geografiche si sono verificate patologie derivanti da malattie epidemiche fino a qualche anno fa del tutto scomparse. Quindi, non sono solo i dati del Ministero della salute alla base del decreto adottato, ma riscontri molto più ampi di soggetti istituzionali diversi, con specifiche competenze e professionalità. Il decreto ora proposto prende atto dell'oggettivo e preoccupante calo della copertura vaccinale - sia pur non trattandosi di emergenza - registratosi negli ultimi anni e della contestuale ricomparsa di alcune malattie da anni dichiarate debellate. In aggiunta, non essendo negli anni scorsi più riscontrabili le patologie debellate o sensibilmente ridotte con le vaccinazioni, è diminuita nella popolazione la percezione dell'importanza delle stesse; ma tali patologie stanno ricomparendo. Secondo i dati del Ministero della salute, è dal 2013 che si registra un progressivo calo della pratica vaccinale, che espone al rischio di focolai epidemici di notevoli dimensioni per malattie attualmente sotto controllo e la ricomparsa di malattie non più presenti nel nostro territorio. Se la media attuale delle vaccinazioni obbligatorie è attorno al 93 per cento, in alcune aree (ad esempio nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Friuli-Venezia Giulia) è addirittura inferiore al 90 per cento. Tra gli ultimi posti figura la Regione Veneto, che nel 2007 ha deciso la non obbligatorietà delle vaccinazioni, attuata a partire da gennaio 2008, e proprio in Veneto, in questa prima parte del 2017, si sono registrati oltre 200 casi di morbillo. Diversità ancora più accentuate si registrano per le vaccinazioni consigliate: a fronte della media nazionale variabile tra l'85 e il 90 per cento a seconda del tipo di vaccinazione, in alcune Regioni o aree geografiche la percentuale è addirittura inferiore al 50 Si riscontra quindi che attualmente le vaccinazioni sono abbondantemente sotto la soglia di sicurezza, in base alla quale il 95 per cento della popolazione dovrebbe sottoporsi a vaccinazione. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha modificato l'assetto dei rapporti istituzionali tra Stato, Regioni ed enti locali, introducendo un quadro di devoluzione delle competenze e delle responsabilità in materia sanitaria. Con questa riforma è stata assegnata alle Regioni la responsabilità, pressoché esclusiva, dell'organizzazione e della gestione del servizio sanitario, mentre allo Stato compete la definizione delle prestazioni sanitarie essenziali (i cosiddetti LEA). Nel panorama sanitario italiano l'offerta di prestazioni vaccinali si presenta attualmente come un mosaico estremamente variegato, con forte eterogeneità territoriale sia a livello regionale (quindi tra Regioni), sia all'interno della stessa Regione, a livello di singole aziende sanitarie Dal punto di vista normativo si sono succeduti provvedimenti che hanno portato ad una progressiva inversione di tendenza sull'obbligatorietà, lasciando ampia discrezionalità alle istituzioni sanitarie locali e ai cittadini. Di fronte ad un problema di questa levatura, un aspetto positivo del decreto-legge è quello di mettere ordine ritornando ad una normativa uniforme a livello nazionale. Da molto tempo la medicina ha individuato nella prevenzione la modalità prioritaria di intervento. Prevenire piuttosto che curare significa intervenire con opportune azioni nei confronti dell'individuo sano per proteggerlo, consentendogli di continuare a vivere bene. questo concetto è stato introdotto con la riforma sanitaria degli anni Ottanta e le vaccinazioni rappresentano sicuramente uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per l'effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati e che non possono essere vaccinati. I vaccini hanno cambiato la storia della medicina e si sono affermati come strumento fondamentale per la riduzione della mortalità e della morbosità, modificando profondamente l'epidemiologia delle malattie infettive.

Dobbiamo allora chiederci il perché del calo della pratica vaccinale. È da ascriversi a cause diverse, *in primis* il diffondersi negli ultimi anni di molti comitati antivaccinali che diramano informazioni generiche, spesso di tipo allarmistico, informazioni non suffragate da adeguate evidenze scientifiche. Si registrano inoltre iniziative da parte di figure istituzionali e professionali che in piena autonomia impartiscono informazioni che si limitano ad evidenziare aspetti negativi (pochi) tralasciando gli indubbi risultati (molti) che la diffusione delle vaccinazioni ha consentito di raggiungere. Non da meno sono i riferimenti a studi e ricerche, smentiti dalla comunità scientifiche, che mettono in relazione vaccinazione ed autismo. Ancora, si è progressivamente diffusa tra i cittadini la falsa informazione che la vaccinazione sia esclusivamente un espediente per arricchire le case farmaceutiche. Altro tema oggetto di grandi discussioni è l'obbligatorietà. Sulla questione dell'ingresso a scuola di bambini non vaccinati si sono sviluppate negli ultimi mesi diverse polemiche, a causa di provvedimenti locali che rischiano di generare ulteriori differenze tra diverse aree geografiche del Paese, oltre a quelle finora provocate dai diversi sistemi di assistenza. Alcune Regioni hanno già introdotto l'obbligo vaccinale per la frequenza degli asili nido. Su tale tema richiamo la sentenza n. 20 del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 16 gennaio 2017, che afferma la legittimità della delibera (tanto criticata) adottata dal Consiglio comunale di Trieste, ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali della fascia da zero «il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale (la libertà dei genitori che ispirandosi ad un principio di precauzione scelgano di non vaccinare i figli) deve regredire rispetto all'interesse pubblico (l'estensione della copertura vaccinale), in particolare dove si tratti di tutela della salute». L'interesse pubblico quindi prevale sulla libera scelta dei singoli. La riduzione e l'eliminazione delle malattie infettive rappresentano una priorità da realizzare attraverso strategie efficaci e omogenee sul territorio nazionale. il 19 gennaio 2017 è stato approvato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il piano nazionale di prevenzione vaccinale, quale strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese. Certamente c'è molto da riprogrammare e da realizzare nel campo dell'informazione, ascoltando attentamente le preoccupazioni dei genitori e lavorando con le comunità e gli operatori sanitari per creare consapevolezza e venire incontro ai bisogni individuali, così che ogni genitore possa assumere decisioni consapevoli per sé e per i propri figli. All'interno del decreto-legge l'esigenza dell'informazione trova risposta nella previsione di un fondo *ad hoc*, anche se ricordo che gli stessi programmi scolastici L'informazione deve essere azione sinergica da attuare con la collaborazione del Sistema sanitario, del personale sanitario, delle istituzioni scolastiche, delle università e dei *mass media*, per favorire e promuovere la cultura vaccinale, mediante l'organizzazione, in maniera ciclica, di incontri con i genitori, convegni tematici, interventi mirati nell'ambito dei corsi di preparazione alla nascita, nei luoghi di lavoro, per informare gli adulti sulle vaccinazioni e sui richiami da effettuare nel corso della propria vita, attraverso l'operato del medico di famiglia, attivando percorsi di informazione permanente. Non va dimenticato che ci sono bambini non vaccinati perché non possono essere vaccinati e che non frequentano la scuola perché rischiano di ammalarsi. Il decreto-legge serve anche per tutelare i diritti di questi e per garantire loro la possibilità della frequenza scolastica. Il decreto-legge tutela quei bambini che, per comprovate motivazioni, rischierebbero conseguenze se vaccinati. In quest'ottica si deve considerare l'introduzione delle sanzioni, peraltro mitigate durante l'*iter* in Commissione. Chiudo questo mio intervento, con il quale intendo esprimere la mia convinta condivisione del decreto-legge, ricordando che in data 18 ottobre dello scorso anno ho presentato come primo firmatario, ad altri componenti del mio Gruppo, una mozione proprio per chiedere quanto viene ora previsto dal decreto-legge; molto di quanto chiesto con quella mozione trova ora risposta in questo decreto-legge.

considerare coloro che sono in piazza come se fossero tutti no-vax o come soggetti che sono lì per difendere la non vaccinazione è un errore. Coloro che sono in piazza fondamentalmente sono lì per chiedere una libera scelta,

Un comportamento di questo tipo rischia di far passare alcuni soggetti dalla categoria dei dubbiosi alla categoria degli scettici, come avevamo detto prima; e questo è molto pericoloso. Paragonare questo anche alla paura per Stamina è un'altra forzatura: su Stamina eravamo tutti d'accordo che fosse una bugia, una truffa, una falsità; sui vaccini, come vedete, c'è un'ampia discussione e non siamo affatto tutti d'accordo, quindi vuol dire, soprattutto sull'obbligatorietà vaccinale, che ci sono dei dubbi. Io cercherò di far capire perché alcuni di noi hanno dei dubbi. Spesso si afferma che coloro che scelgono di non vaccinare i propri figli per motivi di coscienza mettono in pericolo il resto del pubblico e questa è la ragione per porre fine alle esenzioni sui vaccini, attualmente considerate dai legislatori a livello nazionale. Dovremmo però essere consapevoli che la natura della protezione offerta da molti vaccini moderni - e che comprende la maggior parte dei vaccini raccomandati dal CDC (Centers non è coerente con una tale affermazione. Non tutti i vaccini raccomandati possono impedire la trasmissione della malattia o perché non sono progettati per prevenire la trasmissione di infezione (piuttosto, sono sono destinati a prevenire i sintomi della malattia) o perché sono per malattie non trasmissibili. Le persone che non hanno ricevuto i vaccini menzionati di seguito non costituiscono minacce più alte per il pubblico in generale rispetto a coloro che hanno ricevuto la vaccinazione. Ora cercherò di spiegarvi in maniera scientifica il perché. Partiamo dal vaccino del poliovirus inattivato, che non può impedire la trasmissione del poliovirus. Il poliovirus selvaggio è stato assente negli Stati Uniti per almeno due decenni. Anche se il poliovirus selvaggio dovesse essere reimportato in viaggio, il vaccino per la polio con IPV (cioè con il vaccino inattivato) non può pregiudicare la sicurezza degli spazi pubblici. L'eradicazione selvatica del poliovirus è attribuita all'uso di un vaccino diverso, che è l'OPV o vaccino per via orale del poliovirus. Nonostante sia in grado di prevenire la trasmissione selvatica di poliovirus, l'OPV è stato gradualmente eliminato e sostituito con

Il tetano non è una malattia contagiosa, quindi la vaccinazione per il tetano (tramite il vaccino combinato DTaP) non può alterare la sicurezza degli spazi pubblici; esso è destinato a rendere solo una protezione personale. Il vaccino toxoide della difterite, incluso anch'esso nel vaccino difterite-tetano-pertosse, non è stato progettato per prevenire la colonizzazione e la trasmissione di *corynebacterium* *diphtheriae*. La vaccinazione per la difterite non può alterare la sicurezza

che è l'elemento finale del vaccino combinato DTaP, ora in uso, ha sostituito il vaccino della pertosse della cellula intera alla fine degli anni Un esperimento con l'infezione deliberata di pertosse nei primati ha rivelato che il vaccino non è in grado di prevenire la colonizzazione e la trasmissione di *bordetella pertussis.* La pertosse è una malattia respiratoria altamente contagiosa: i tassi di pertosse negli Stati Uniti sono aumentati e hanno raggiunto i 42.000 casi nel 2012. Sebbene la rinascita della pertosse non sia completamente compresa, ipotizziamo che i vaccini pertussici acellulari, contenuti nel vaccino trivalente, non riescono a prevenire la colonizzazione e la trasmissione. I babbuini vaccinati con tale vaccino sono stati protetti da gravi sintomi associati alla pertosse, ma non dalla colonizzazione e hanno subito trasmesso la *bordetella pertussis* a contatti non vaccinati. Per confronto, gli animali precedentemente infetti non sono stati colonizzati per infezione secondaria. Quindi, il controllo ottimale della pertosse richiederà lo sviluppo di vaccini migliorati. Facciamo pertanto la ricerca in questa direzione. Inoltre, la riunione del consiglio dei consiglieri scientifici del CDC del 2013 ha rilevato che le persone vaccinate per la pertosse hanno più probabilità di essere infetti e quindi contagiosi rispetto alle persone che non sono vaccinate. Veniamo ai numerosi tipi di *haemophilus influenzae*. Il vaccino *haemophilus influenzae* B copre solo il tipo B. L'introduzione di questo vaccino ha inavvertitamente spostato la dominanza del ceppo verso altri tipi di *haemophilus influenzae*, cioè quelli che vanno dalla La popolazione generale è vulnerabile alla malattia invasiva più di quanto non fosse prima dell'inizio della campagna di vaccinazione per l'Hib. La discriminazione contro i bambini bambini non vaccinati per Hib, quindi, non ha alcun senso scientifico nell'era della malattia *haemophilus influenzae* di tipo h.

Quindi, i bambini vaccinati per l'epatite b non possono alterare in alcun modo significativo la sicurezza degli spazi pubblici. Inoltre, l'ammissione alla scuola non è proibita per i bambini portatori di epatite b cronica. vietare l'ammissione a scuola a coloro che sono semplicemente non vaccinati e non portatori di epatite b costituirebbe una discriminazione di tipo irragionevole e illogico. Veniamo ora al morbillo. cito l'articolo di Poland e Jacobson del 1994, in cui si sostiene che il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione del morbillo è un paradosso apparente delle infezioni da morbillo nelle persone immuni. Il paradosso apparente è che quando i tassi di immunizzazione del morbillo aumentano ad alti livelli in una popolazione, il morbillo diventa una malattia di persone immunizzate. Ulteriori ricerche hanno determinato che dietro il paradosso del morbillo vi è una frazione della popolazione chiamata basso *responder* di vaccino. I pazienti con bassa risposta sono coloro che rispondono male alla prima dose del vaccino contro il morbillo. Questi individui montano una debole risposta immunitaria alla successiva vaccinazione e ritornano rapidamente alla piscina di suscettibili entro due-cinque anni, nonostante siano stati completamente vaccinati. La rivaccinazione non riesce a correggere una scarsa risposta, che sembra essere un tratto immunogenico. Gli studi sull'epidemia di morbillo in Québec (Canada) e Cina attestano che persistono focolai di morbillo anche quando la conformità alle vaccinazioni è alla massima clausola, ossia 95-97 per cento, e persino al 99 Ciò è dovuto al fatto che anche nei pazienti con elevata risposta al vaccino gli anticorpi indotti dal vaccino sono diminuiti nel tempo. A questo punto, veniamo alle considerazioni sulla sentenza della Corte di che stabilisce un principio che farà giurisprudenza in tutta l'Unione europea. Nella sentenza si statuisce che non è necessaria la prova medico-scientifica per stabilire un nesso tra la somministrazione di un vaccino e la malattia che colpisce in seguito un paziente, essendo sufficienti indizi purché siano «gravi, precisi e concordanti». Si tratta di un verdetto che permetterà a molti pazienti di intentare causa contro le case farmaceutiche. In pratica, non serve più la prova certa che la patologia sia causata direttamente dalla somministrazione del vaccino. Sono considerati indizi sufficienti da parte del giudice il fatto che la malattia sia insorta a poca distanza dalla vaccinazione e l'assenza di precedenti medici personali o familiari. Quindi, inserire l'obbligatorietà vaccinale da zero a sedici anni per 10 o 12 vaccinazioni con molta probabilità aprirà la strada a numerosi contenziosi di tipo risarcitorio. C'è da dire un'altra cosa per me fondamentale, in quanto medico. Questo provvedimento coercitivo mina profondamente il rapporto tra medico e paziente,

Le motivazioni che spesso inducono i genitori a ritardare le vaccinazioni o a non vaccinare indicano spesso nell'età troppo precoce del bambino la causa principale, considerando questa età come vulnerabile e troppo suscettibile agli eventi avversi. Un'altra causa importante è la mancata comunicazione oppure una comunicazione troppo superficiale da parte degli operatori sanitari dei centri vaccinali, che fanno riferimento solo ai vantaggi e non parlano mai dei possibili rischi avversi. Tutto questo aumenta la diffidenza da parte dei genitori. Infine la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini ad una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse che, secondo l'AIFA, solo nel 2013, per l'esavalente sono stati 1.343 di cui 141 gravi. È utile rammentare che le reazioni avverse ai farmaci (non solo ai vaccini) sono state indicate nel 2008 come la quinta maggiore causa di mortalità ospedaliera in Europa. Resta l'impossibilità, poi, di ricorrere a vaccini in forma singola e l'indisponibilità sul mercato dell'antidifterico se non abbinato ad altri vaccini.

Risulta quindi evidente, da tutto quello che ho detto, che l'unica vera base scientifica che è presente in questo decreto-legge è che scientificamente, visto che non esiste al momento alcuna precedente ricerca sulla somministrazione di 10 o 12 vaccinazioni obbligatorie per tutti i soggetti non vaccinati nella fascia di età zero-sedici anni, il Ministero della salute, in accordo con l'Istituto superiore di sanità (o viceversa), ha deciso di fare un sperimentazione di massa su tutti i bambini italiani e, alla fine di questa sperimentazione, ci daranno i dati scientifici solidi, con i numeri precisi di eradicazione eventuale di malattie contagiose e quanto questo è costato in termini di eventi avversi più o meno gravi. Prima della fine di questa sperimentazione non possiamo avere risposte certe ad alcuna di queste domande, perché, scientificamente parlando, è alla fine che avremo la risposta; prima siamo nel campo delle ipotesi da verificare attraverso la ricerca. Io, come essere umano, non mi considero un mezzo per la realizzazione di un processo sanitario ma il fine. ma il fine. Purtroppo tutte le reazioni *post*-vaccinali vengono negate, in quanto dovute a sfortunate coincidenze. In Giappone quando hanno spostato le vaccinazioni a due anni si sono ridotte notevolmente le morti in culla. Può essere un caso, forse, non lo so. L'esavalente è approvato fino a trentasei quindi se lo rendiamo obbligatorio fino a sedici anni non abbiamo alcuna sperimentazione. A questo punto vi spiego perché non sono un no vax. Perché una parte consistente di chi si dichiara no vax è alleato con - e a volte utilizzato da - quel bacino di cittadini o di popolo che vedono nello Stato un nemico da abbattere, una realtà ostile da cui difendersi. In tutto questo i bambini sono diventati il campo di battaglia: «Giù le mani dai nostri figli», come è già successo al Family day. L'anti-Stato fa parte della storia d'Italia ed ora è la volta dei genitori, tutto questo scatenato dalle pretese di un controllo totale da parte dello Stato e, dall'altro lato, una pretesa uguale da parte delle famiglie. Ecco che lo Stato è visto come un'autorità da cui difendersi, quando il nostro compito dovrebbe essere quello di renderlo una realtà cui tutti partecipano. Non agire in questa direzione porta solamente alla vittoria delle piccole identità, delle piccole comunità, contro la grande comunità dello Stato. Il vero paradosso è che sono costretto a parlare di questo, non per giustificare i giusti interventi a favore di una comunità economica e sociale, ma per una comunità di tipo sanitario. In pratica, lo Stato interviene perché una società non vaccinata è pericolosa. Se ci limitiamo a questa affermazione però non sapremo qual è il livello del pericolo e quali sono le strategie da mettere in atto per ridurre o eliminare questo pericolo; meglio ancora se queste strategie vengono condivise e non risultino impositive. Ho sentito molte volte parlare il Ministro e il direttore dell'Istituto superiore di sanità di un bellissimo esempio dato dal governatore della California per alzare il livello di copertura vaccinale per il morbillo di 5 punti percentuali in due anni, attraverso l'obbligatorietà vaccinale. A parte la mancanza di dati scientifici a sostegno di questa tesi (e ciò di per sé è già grave), forse ci siamo dimenticati che stiamo parlando della Nazione che più di tutte le altre è fondata su una ontologica diffidenza verso lo Stato e sul diritto costituzionale dei suoi cittadini a ribellarsi all'autorità centrale. Siamo quindi di fronte ad una Nazione la cui base filosofica si basa sul principio della sfiducia nei confronti dello Stato - ciò è molto diverso dal nostro modo di pensare - e anche nella sfiducia verso le case farmaceutiche, che in America hanno falsificato i dati clinici sull'affidabilità degli oppioidi nella terapia del dolore. truffa è alla base dell'abuso di tali sostanze, con il conseguente aumento di decessi da overdose negli Stati Uniti: oltre 60.000 nel 2016. Non dimentichiamo, infine, che il cospirazionismo è l'altra faccia, deformata, di una sana diffidenza nei confronti dello Stato. Per finire, Per finire, come non ricordare in questo percorso le perle del professor Burioni, che insulta le persone sul suo profilo Facebook e su Twitter e che viene acclamato da esponenti del Governo

Cito un'altra perla di saggezza: «Siete solo un branco di somari raglianti. Facebook vi ha illuso di contare qualche cosa con la vostra mente atrofizzata e con il vostro italiano claudicante. Invece non contate nulla, dovete solo essere messi in condizione di non nuocere.» - e non oso pensare come - «La scienza non è democratica». A questo punto mi spiace dirvelo, ma se vi fidate ciecamente - anzi, direi come professione di fede - della scienza di tali scienziati, avete veramente un serio problema.

Signora Presidente, intervengo per sollecitare l'attenzione dell'Assemblea sui gravissimi roghi che da diversi giorni stanno flagellando il Vesuvio. La situazione è molto più drammatica di come probabilmente è stata percepita dagli organi che avrebbero dovuto intervenire immediatamente, ma che lo hanno fatto con un certo ritardo. Il Vesuvio brucia, a causa di otto incendi innescati in otto punti diversi. Addirittura si ipotizza l'uso di animali vivi utilizzati come esche per alimentare ulteriormente l'incendio.

famiglie evacuate, tensione e fumo nero, denso e irrespirabile: una colonna immensa, tragica, colma di cenere, che si posa sulle città vesuviane nell'indifferenza di chi, anche in quest'Aula, non ha voluto ascoltare il grido di allarme quando abbiamo discusso della legge delega sulla protezione civile e ancora ci sembra poco attento alla tragedia immane che stanno vivendo le popolazioni vesuviane. la paura che le fiamme possano raggiungere le discariche e moltissimi rifiuti abbandonati in tante aree private e parliamo di zone come Ercolano, la città degli scavi, e Terzigno, altra città bellissima. Sono posti straordinariamente belli e incantevoli che si stanno distruggendo a causa di questi feroci e tragici roghi. Mi chiedo e le chiedo, signora Presidente, in rappresentanza del Senato: è stata una scelta giusta quelli di accorpare il Corpo forestale dello Stato ai Carabinieri,

È stata una scelta giusta quella di non potenziare, di anno in anno, la flotta aerea di Canadair e di attrezzature antincendio? Siamo sicuri che l'affidamento dei compiti di protezione civile alle Regioni sia la soluzione giusta? Il piano delle attività antincendio boschivo, che è stato emanato con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio, è stato oggettivamente disatteso, altrimenti non ci troveremmo di fronte a una simile tragedia e agli Continuare a ritenere che i sindaci siano autorità di protezione civile è un sistema fuorviante per rappresentare ai cittadini il modo di fare le leggi che vige nel nostro Parlamento.

Se invece continuiamo con questo articolato di norme, nel quale nessuno sa esattamente cosa fare quando succedono queste tragedie, ci troveremo purtroppo sempre più a nutrire

si verificava la collisione fra due treni della compagnia ferroviaria Ferrotramviaria. Un incidente in cui hanno perso la vita 23 persone, fra le quali i macchinisti di entrambi i convogli e un capotreno, e circa 50 persone sono rimaste ferite. Si tratta del più grave disastro ferroviario mai avvenuto sul territorio pugliese, uno dei più drammatici incidenti registrati nel nostro Paese. Siamo rimasti tutti sconvolti di fronte alle immagini di quelle lamiere contorte fra gli ulivi. In silenzio abbiamo seguito, attraverso gli organi di informazione, le difficili operazioni di soccorso e di intervento. È stato un lutto collettivo e nazionale, che oggi vogliamo ricordare anche in segno di vicinanza alle tante famiglie che soffrono per questa ricorrenza, rispetto alla quale ogni parola appare, sebbene sentita e spontanea, comunque superflua, perché di fronte al dolore della perdita ogni parola rischia di essere tale. I treni stavano viaggiando in direzioni opposte. La presenza di una curva non ha consentito ai macchinisti alcuna possibilità di avvistamento e non è stata possibile alcuna frenata di emergenza. Su quella tratta a binario unico, dove era operativo il solo sistema del blocco telefonico, non è stato dunque possibile evitare l'impatto. La Procura di Trani ha aperto un'indagine ipotizzando i reati di disastro ferroviario ed omicidio colposo plurimo. Come Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta il fenomeno degli infortuni sul lavoro, ho promosso l'apertura di un'indagine e lo scorso 22 luglio, appena dieci giorni dopo la tragedia, ci siamo recati, assieme al collega Daniele Borioli e alla senatrice Pelino, sul luogo del disastro ferroviario. Sono immagini, Presidente che non possiamo dimenticare, così come non possiamo dimenticare la richiesta di verità e giustizia che proviene dalle famiglie delle vittime, cui, come Stato e come istituzioni, abbiamo il dovere di dare risposta. Attendendo l'esito del lavoro, indefesso e serio, che sta portando avanti la Procura di Trani, abbiamo chiuso, per quanto è di nostra competenza, l'indagine della Commissione, i cui risultati renderemo noti entro la fine di questo mese. È il nostro contributo all'esigenza di chiarezza, di verità e di giustizia che dobbiamo alle vittime, ai loro cari, ma anche a tutte le cittadine e tutti i cittadini. La sicurezza, signora Presidente, è un tema cui non possiamo e non dobbiamo venir meno, perché il dolore che abbiamo provato in occasione di quel tragico incidente non si trasformi, in occasione di ogni anniversario, in una retorica commemorazione, ma sia invece motore non solo della ricerca della verità ma anche dell'impegno per la prevenzione. Signora Presidente, attualmente l'industria del cinema è ferma. I lavoratori del cinema stanno a casa, i produttori non girano. Nel novembre 2016 è stata approvata, con squilli di tromba, una nuova legge sul cinema: Renzi e Franceschini ricevono grandi autori, registi, attori - tutti sostenitori del sì al *referendum* - convinti che l'ex *Premier* avrebbe rilanciato l'industria con 400 milioni di euro. La legge prevedeva che la fetta più grossa fosse per i grandi produttori inseriva automatismi che favorivano chi otteneva risultati economici e artistici rilevanti. Ad oggi è tutto fermo, non si lavora e non si produce. Perché? motivo è che si è pasticciato con le norme della legge di stabilità del 2015. Parliamo, quindi, di molto tempo fa. E già nel 2016 si è quasi bloccato tutto il settore perché mancavano i decreti attuativi. dopo l'approvazione della legge sul cinema, il film non è cambiato. La storia è rimasta la stessa: continuano a bloccare tutto mancando i decreti attuativi. è andata in onda la famosa puntata di «Report» e scopriamo che il problema non sono solo i benedetti decreti attuativi ma anche i potenziali illeciti

il Ministero e i piccoli produttori. Perché anche i piccoli produttori chiedono che i decreti attuativi siano equi e che, giustamente, rispettino anche loro e non solo Anica nella definizione delle norme e degli automatismi per l'erogazione dei fondi del *tax credit*. Quindi, io chiedo al Governo che si dia una mossa perché davvero la situazione è drammatica. Mibact e Mise devono fare i decreti attuativi, altrimenti quest'anno, fino a fine 2017 e oltre, il settore resterà bloccato e i lavoratori staranno a casa.

Presidente, intervengo nuovamente in questa Aula per sollecitare la nomina dei senatori che devono comporre la Commissione monocamerale d'inchiesta sulla ricostruzione *post*-sisma dell'Aquila. Lo faccio per l'ennesima volta, e lo farò ogni settimana fino quando non si procederà alla sua effettiva composizione. Lo scorso 28 giugno, dopo il mio intervento di fine seduta, il presidente Grasso aveva assicurato che «la Presidenza ha già sollecitato e solleciterà ancora una volta i due soli Gruppi che non hanno presentato le designazioni» e che «sarà cura della Presidenza cercare di acquisire tutte le designazioni». Due Gruppi parlamentari non hanno, quindi, ancora designato i senatori che dovrebbero far parte della Commissione d'inchiesta e con la loro condotta hanno di fatto, fino a questo momento, impedito che la Commissione d'inchiesta sia già operativa. Forse - e mi rivolgo anche in questo caso direttamente alla Presidenza - sarebbe importante sapere quali siano i due Gruppi che non vogliono si faccia chiarezza sulle responsabilità politiche nazionali e locali in merito ad alcune vicende poco trasparenti legate all'utilizzo dei fondi per la ricostruzione. E ne è una testimonianza lo stato di fatto della città città dell'Aquila e dei crateri. Ricordo ancora una volta alla Presidenza che la Commissione d'inchiesta è stata deliberata da quest'Assemblea il 10 novembre scorso, con l'approvazione del relativo documento a mia prima firma. Da allora è trascorso un lasso di tempo molto ampio che avrebbe permesso di svolgere un lavoro incisivo. Con il mio intervento, pertanto, le chiedo, signora Presidente, ai sensi dell'articolo 2, del documento che istituisce la Commissione d'inchiesta, di procedere il prima possibile alla nomina dei componenti, sollecitando ancora una volta i Gruppi parlamentari

e soprattutto i due Gruppi parlamentari - che finora hanno di fatto impedito l'avvio di questa importante Commissione d'inchiesta. Avviamo rapidamente i lavori:

delicatissima di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani: una questione inerente alla discussione, che oggi abbiamo avuto in Assemblea, sui vaccini.

di grande cuore, sensibilissima, affinché possa riportare al presidente Grasso il dubbio che tutti abbiamo nel nostro cuore e nella nostra testa su un fatto importantissimo, che vorremmo capire prima di votare. Lei sa meglio di me,

era accertato, cioè, un conflitto di interessi per questo signore che si chiama Pecorelli e che oggi è uno dei due che redigono il piano vaccinale a livello nazionale. Mi rivolgo a lei, Presidente, perché non so a chi rivolgermi: ho grande confusione, non capisco più niente, ho difficoltà a capire come italiano quale sia la verità: la verità: qualcuno mi dice che sono importantissimi 12 vaccini, poi scendiamo a 10 (quindi, due non erano importanti). Un piano che non si riesce a capire da dove entra e da dove esce; che viene definito urgentissimo ma poi all'ultimo momento si può fare anche mediazione politica. Mi rivolgo a lei, allora, con il cuore in mano, da padre di famiglia

per arricchire le *lobby* farmaceutiche e per danneggiare suo figlio, Presidente, mio figlio e il figlio di coloro i quali non la pensano come me ma chi è il figlio di un padre e di una madre. Noi parlamentari abbiamo l'obbligo di difendere gli italiani… sta facendo un intervento che non dovrebbe fare. tutti all'interno di quest'Aula parlamentare e fuori di essa, chi pro e chi pronto, tentiamo di fare gli interessi dei nostri figli, dei figli dei nostri amici ed anche di coloro i quali non sono amici. Presidente, la